che sia chiaro che sia stata posta la questione di fiducia in modo corretto. Noi abbiamo sentito l'audio e c'è un passaggio in cui si sta per fare questa dichiarazione, ma il presidente

Da questo punto di vista, il verbale può essere posto in votazione, ma solo ed esclusivamente quando ci siano delle difformità rispetto alle parti politiche, non quando esso non rispecchia la realtà dei fatti, perché sulla realtà dei fatti l'autorità è quella del Presidente del Senato. Noi non riteniamo dunque che ci siano le condizioni per procedere alla votazione del processo verbale anche perché, se così fosse, avremmo poi il problema di cosa scrivere in luogo di quello che è stato votato

Capigruppo con una decisione sul calendario che mi pare condivisa: non l'abbiamo votata, quindi c'è stata una decisione sul calendario condivisa. Ciò vuol dire che tutti

presidente La Russa, nella riunione dei Capigruppo, ha attestato il fatto che il ministro D'Incà aveva

insensata e trovo anche insensato votare un verbale che non fa altro che riconoscere ciò che ieri è successo, cioè che ieri è iniziata la discussione sulla fiducia.

nella prima riunione, ma per la verità precisando ancor di più avendo controllato bene il verbale,

correttamente posta la questione di fiducia, peraltro asseverata anche dallo stesso vice presidente La Russa che presiedeva. Il presidente Romeo era presente alla riunione dei Capigruppo e lo sa perfettamente.

stenografico. Si può chiedere di mettere in votazione il verbale perché si vuole aggiungere una precisazione, ma tutta la discussione di ieri, anche formalmente, nella riunione dei Capigruppo si è magari soffermata sulle modalità, sul fatto se si sgombrava l'Aula o no, se si iniziava la discussione generale ieri sera o questa mattina, ma quel presupposto non è stato messo in discussione. Non so se la notte ha modificato i dati

di parlare per mettere la fiducia, questo l'abbiamo capito, ma siccome questo è avvenuto e la fiducia è stata posta correttamente, credo che oggi si possa far aggiungere qualsiasi cosa al verbale, ma non certamente mettere in discussione, attraverso la votazione su quel punto, il fatto che il Governo abbia correttamente posto la questione di fiducia, leggendo il verbale, leggendo il dispositivo e dicendo con chiarezza che la fiducia veniva posta sul testo del decreto trasmesso dalla Camera. Signor Presidente, a fronte di questi argomenti è sempre meglio prendere in mano il Regolamento. È evidente che la proposta che ha fatto il presidente Romeo non ha alcunché di ostruzionistico, perché il nuovo Regolamento non prevede, non prevede, per la votazione del processo verbale, neppure la verifica del numero legale, come accadeva un tempo. La proposta pertanto non ha, quindi, un significato ostruzionistico, ma un significato politico e di verità. Leggo cosa dice l'articolo 60 del Regolamento: «Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato». Se si deve procedere alla votazione, questa si fa per alzata di mano e non deve essere chiesto il numero legale. Quello che contesta il presidente Romeo, e che io condivido...

commettevano un illecito. Il presidente Romeo dice: io non riconosco il fatto di cui è stato dato lettura, ovvero l'apposizione della questione di fiducia. Quando questo è accaduto, mi trovavo a fianco dello scranno del Presidente perché avrei dovuto subentrare al presidente La Russa. Da quella posizione, quindi immediatamente dietro la posizione in cui era il ministro D'Incà, io le dico che ho sentito le prime due o tre parole che ha detto il ministro D'Incà e le successive non sono riuscito. Però, causa la mia alta età (probabilmente soffro di ipoacusia), ipoacusia), sono andato a sentirmi per dieci volte l'audio, che è consultabile sul sito del Senato. E ancora dopo averlo sentito dieci volte, quella frase che ritrovo nel resoconto stenografico non l'ho riscontrata. Sarà un problema mio? Sono sordo? Va bene, ma anche altri evidentemente non l'hanno sentito. Visto che invece, evidentemente, abbiamo qualcuno che è dotato di uno sviluppo dell'udito così eccezionale da riuscire a mettere gli articoli, i numeri, il giorno e la data, mi complimento. Io non mi sento di votare a favore di un resoconto stenografico che, senatore Licheri, è un falso in atto pubblico quando dovesse essere approvato. Fintanto che non è ancora approvato, non c'è nessun falso in atto pubblico. Il voto che noi chiediamo è un'azione preventiva rispetto al fatto che si crei il presupposto del reato, cioè del falso in atto pubblico.

non è che si chiude la seduta e non si può procedere. Quindi non capisco il perché di questi continui interventi *(Applausi)*, che mi fanno pensare a un ostruzionismo di maggioranza a questo punto.

Intanto sono esauriti gli interventi, perché la parola, ai sensi del comma 3 dell'articolo 60, è concessa solo a chi intenda farvi inserire una rettifica, per fatto personale o per semplice annuncio di voto.

del verbale per alzata di mano, con procedimento elettronico dato il carico che ci siamo fatti di chi non può stare in Aula. rettificare il verbale voterà sì, chi non intende rettificare il verbale voterà no. La rettifica La rettifica è quella che è stata proposta dal presidente Romeo. È una sola. La votazione è aperta.

Colleghi, consentite a tutti di votare, come abbiamo sempre fatto quando c'è una prima votazione. Questo vale assolutamente per tutti.

io non chiudo la votazione finché tutti non prendono il proprio posto e non cessano le intemperanze in Aula.

Siccome non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato così come ne è stata data lettura. apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina

consideriamo che nella giornata di ieri già si sono verificati alcuni fatti di intemperanza e abbiamo giustamente

dunque tutta l'Assemblea ad osservare un comportamento conseguente e degno, anche perché non c'è motivo

al modello decreto tarocco. L'urgenza di emanare il decreto-legge in esame è contenuta solamente nel titolo. In Italia, dal 31 gennaio è stato dichiarato lo stato di emergenza per motivi di salute pubblica, stato prorogato fino al 31 gennaio 2021. Dai primi di marzo gli italiani hanno iniziato a lottare per sopravvivere al Covid-19, da un lato, e alla crisi economica, dall'altro. Nel mentre, attraverso diversi DPCM, si sono visti limitare e in alcuni casi sospendere molti dei loro diritti. Hanno accettato questa privazione, dimostrando senso di responsabilità e rispetto delle regole. Ebbene, se qualche italiano trovasse il tempo di leggere le 251 pagine del decreto-legge in esame, si renderebbe conto che non c'è un solo articolo che interviene su situazioni emergenziali. Inoltre si renderebbe conto del paradosso delle decisioni del Governo, che da una parte chiude i porti alle navi da crociera, nonostante si fossero adoperate per adeguarsi alle misure anticontagio, operando così in sicurezza, ma li mantiene spalancati per chi decide di approdare, senza chiedere autorizzazione e senza la minima misura di prevenzione anti-Covid. Proprio in tal senso, viene da chiedersi - anzi, lo chiedo al Governo - che fine ha fatto il decreto interministeriale del 7

con la conseguenza di non poter acconsentire agli sbarchi. Chiedo al Governo che fine ha fatto questo decreto: se esiste ed è ancora in vita, oppure se è stato abolito.

Quale futuro riuscite a garantire alle persone che sono arrivate, quando non siete neanche in grado di garantire il presente agli italiani? futuro cui li destinate assomiglia alla situazione che troviamo davanti alla stazione di Roma Termini, dove uomini e donne bivaccano giorno e notte, espletando i loro bisogni accanto a dove dormono, senza una meta e private della loro dignità. Questo è quello che riguarda il futuro. Per quanto riguarda

Ebbene, lì non esiste distanziamento e ci sono uomini, donne, bambini e minori non accompagnati in situazione di promiscuità

Ma voi siete quelli buoni, quelli del «restiamo umani». Questo è il vostro modo di gestire l'immigrazione. Questo è quello che avete sempre fatto: lanciare messaggi illusori che portano migliaia di persone ad arrivare in Italia per poi scaricare il problema sulla società. *(Applausi)*. Illudete i ragazzini, inducendoli a lasciare la propria famiglia e i propri cari, nella speranza di trovare chissà quale prospettiva di futuro qui da noi. Quando al Ministero dell'interno c'era quel cattivone di Salvini non ci sono stati morti a bordo delle navi, in quanto donne, bambini e persone che avevano bisogno di cure sono sempre stati fatti sbarcare.

la cui morte non ha fatto scalpore; magari, forse, meno se ne parla e meglio è, perché qualcuno ha delle responsabilità e c'è un'inchiesta aperta. Però noi eravamo quelli cattivi e voi siete quelli buoni...

La cosa che più mi dispiace e un po' mi stupisce - ma, dopo sabato, il mio stupore è venuto meno - è che una parte della maggioranza attuale

territorio e tradizioni. Voglio citare il mio bellissimo Comune, Fiumicino: la nostra amministrazione ha concesso l'opportunità di realizzare i canti natalizi, ma senza riferimenti religiosi. Ora in Italia ci dobbiamo vergognare di essere cristiani? No, non ci vergogniamo di essere cristiani: rivendichiamo la nostra appartenenza culturale e religiosa. Quanto l'Italia ha dei confini e la Costituzione, insieme alle leggi internazionali, ci impongono il controllo, sia materiale che militare, dei nostri confini. Ricordiamolo: siamo una Nazione che deve difendere i propri confini, perché noi qui siamo senatori della Repubblica italiana e dobbiamo tutelare gli interessi degli italiani, e non gli interessi di cittadini di altre Nazioni. Siamo orgogliosamente italiani.

A tutti gli altri cittadini di altre Nazioni non è concessa la libera circolazione nella nostra Nazione e nemmeno in Europa. Quando parliamo di

altrimenti si favorisce un'immigrazione che produce non integrazione, ma emarginazione e delinquenza. Ma che cosa vi hanno fatto gli italiani per trasformare le nostre città e le nostre periferie in zone di degrado, i nostri parchi in zone di spaccio di immigrati irregolari? Che cosa vi hanno fatto di male gli italiani, che li state tradendo tutti i giorni? In più, signori miei, vorrei stendere un velo pietoso su una storia che ci ha visto tutti coinvolti, ad applaudire da una parte e a contestare dall'altra: la signora Rackete che ha volontariamente investito un'imbarcazione militare della Guardia di finanza, un'eroina per la sinistra che è stata tre giorni agli arresti domiciliari. A Firenze dei ragazzi, non di sinistra, che hanno fatto un volantinaggio non autorizzato sono da quattro settimane agli arresti domiciliari, perché non sono di sinistra. Vergogna! *(Applausi)*. Non cederemo alle vostre pressioni. Non cederemo alle vostre intimidazioni. Non tradiremo i figli d'Italia. Non tradiremo la nostra Nazione, per un semplice motivo: non ci arrenderemo mai, ma continueremo la nostra battaglia per il nostro più grande amore, ossia la nostra amata Italia.

i decreti sicurezza voluti da Matteo Salvini, che erano stati adottati per venire incontro alle legittime istanze degli amministratori locali, delle Forze dell'ordine e degli stessi cittadini. Questo decreto-legge, invece, ha avuto come interlocuzione solo le ONG. infatti, ampliata la disciplina dei permessi di soggiorno e di altri titoli di soggiorno analoghi, la disciplina della protezione internazionale, la disciplina del trattenimento degli stranieri ed è stata completamente modificata la disciplina dei divieti all'ingresso di navi nel mare territoriale e delle relative sanzioni. la disciplina dei termini relativi ai procedimenti in materia di cittadinanza e quella relativa alle funzioni, agli *standard* di servizio e alle tipologie di prestazioni, nonché ai beneficiari del sistema di accoglienza. Per evitare quindi un'accoglienza indiscriminata la Lega ha proposto, sia alla Camera che al Senato, una serie di emendamenti, che non ci avete consentito di discutere, al fine di poter dare un contributo costruttivo e non ostruzionistico e di aiutare e collaborare con i nostri amministratori locali con le nostre Forze di polizia. Noi della Lega abbiamo proposto una collaborazione leale - un termine sconosciuto ormai a questa maggioranza *(Applausi)* - tra i livelli di Governo interessati, all'interno dei quali coesistono strutture di vario tipo e differenti funzioni. Invece non è stato così. Ricordo che la disciplina precedente rispetto ai decreti Salvini consentiva a tutti i prefetti di distribuire i migranti senza informare preventivamente gli amministratori locali o informandoli solo nell'imminenza degli arrivi. Da parte di quel Governo a firma PD vi era un certo abuso di potere. In quel periodo sono state moltissime le manifestazioni spontanee delle comunità locali che, assieme ai propri sindaci, hanno protestato contro l'ingresso nel proprio territorio degli immigrati. Con questo provvedimento ritorneremo a quel periodo, signor Presidente, perché le responsabilità nella gestione dell'emergenza migratoria ricadranno inevitabilmente sugli enti e sulle comunità locali per paura di essere rimossi, saranno costretti a eseguire le direttive del Ministro dell'interno in tema di distribuzione di migranti, senza avere alcuna possibilità di consultare i sindaci, come già avveniva con quei precedenti Governi di centrosinistra. riduce le possibilità di intervento di sindaci e amministratori locali, con il rischio che essi possano trovarsi a gestire situazioni molto delicate sul piano dell'ordine pubblico. *(Applausi)*. È per questo che avevamo proposto una serie di emendamenti riferiti alla polizia locale - tutti chiaramente chiaramente non discussi - in considerazione del fatto che questo provvedimento rafforza alcune misure in materia di divieto di accesso a locali ed esercizi pubblici, la cui applicazione dovrà essere garantita proprio dalla stessa. L'arrivo e la permanenza continuativa di un elevato numero di migranti, le ulteriori misure in materia di divieto e di accesso a servizi e locali pubblici, la cui applicazione è rimessa in buona parte alla polizia locale, accresceranno verosimilmente la percezione di insicurezza nel nostro Paese in questo momento. Comunque, signor Presidente, con questo decreto-legge noi oggi assistiamo a un cambio di passo vero: vero: tutela ai clandestini e meno tutela ai diritti degli italiani. Ormai è chiaro che questo Governo crea delle disuguaglianze sociali vere, così come è evidente che è formato da un *mix* di forze politiche e non pensa agli italiani

Oggi non lo sappiamo, ma presumiamo dalle indiscrezioni che ci sarà una chiusura totale. Non sarebbe male saperlo prima, perché ognuno deve anche farsi dei programmi, specialmente se deve fare dei viaggi. Chi ha ristoranti e aspetta da mesi questo momento, che rappresenta una percentuale importante del proprio fatturato, ha fatto delle scorte e ha comprato degli alimenti, i quali non sono come i DPCM che, finito uno, ne fai un altro a costo zero per chi lo firma.

facile e più difficile il contrasto all'immigrazione clandestina. Questo è un fatto chiaro, è scritto in ogni parte del decreto-legge, e su questo il Governo ha pensato per tempo, perché è un decreto di ottobre.

vincola, sia pure in modo non assoluto, i senatori della maggioranza. Riguardo all'immigrazione, prima di pensare ad allargare le maglie, in modo da rendere più difficile il contrasto all'immigrazione clandestina, le leggi

del tutto diversi e, proprio per questo, andrebbe gestita in modo ordinato. Pensare di azzerarla è impossibile, ma anche pensare di aprire le porte, più o meno indiscriminatamente, a chi entra illegalmente è estremamente negativo. Sappiamo tutti che sono moltissimi gli stranieri molto bene inseriti nella nostra società. Certi settori avrebbero difficoltà a andare avanti senza degli stranieri,

il nostro Paese. La preoccupazione dovrebbe essere come far rispettare le leggi. Chi vuole immigrare legalmente nel nostro Paese incontra degli ostacoli enormi, senza fine, con pratiche che durano anni. Persone, che sono qui da

spezza la vita a chi li utilizza. Ecco, si rende la vita più facile a quelle persone. Francamente, non credo davvero che questa fosse una priorità.

La prova delle difficoltà di inserimento di quelle persone nel nostro Paese c'è anche senza andare a spizzicare nella cronaca: basta leggere i dati e le statistiche, quelle ufficiali, dell'Istat e del Ministero della giustizia.

del femminicidio e la settimana dopo dell'immigrazione, non integrando le questioni, vuol dire che si avanti a *spot*, si va avanti per ideologia, si va avanti per tentare di fare il titolo e compiacere questo o quel gruppo di influenza.

più difficili e in continua evoluzione, all'incirca il 50 per cento di coloro che sono negli istituti penali minorili. È evidente che c'è un gravissimo problema di inserimento e che, con

Qual è l'urgenza per la maggioranza? Aumentare ulteriormente l'immigrazione clandestina. È veramente una cosa difficile da comprendere, se non con un approccio ideologico. Quando però l'approccio ideologico è alternante, la cosa diventa ancora più preoccupante. I colleghi del MoVimento 5 Stelle si apprestano a votare la cancellazione di norme che hanno approvato meno di due anni fa, durante il primo Governo Conte, e che adesso per motivi ideologici cancellano. Francamente credo che molti di loro siano in imbarazzo. Penso che la maggior parte di loro siano persone che hanno intrapreso l'impegno politico

ricevevano regolarmente i complimenti dai colleghi del MoVimento 5 Stelle che volevano differenziarsi da noi di Forza Italia che avevamo richiesto questa indagine e dagli altri colleghi del centrodestra che la portavano avanti.

invece, di aumentare l'immigrazione clandestina. Non stupitevi se poi lo sdegno si manifesta in vari modi, a volte anche non condivisibili, ma di certo non è la strada giusta quella che state prendendo. Signor Presidente, con il provvedimento in esame oggi continuiamo una discussione che ha rasentato veramente il surreale sia in Commissione, sia in Aula. Sul metodo di lavoro penso che non ci sia nemmeno da spendere parole, visto che i fatti hanno dimostrato in questi giorni come su un decreto-legge su una materia così importante come l'immigrazione, che non è - con tutto il rispetto - il codice della strada, ci troviamo a discutere e a non discutere, con mortificazione del dibattito, addirittura con l'eliminazione degli spazi che potevamo avere anche per fare delle proposte emendative. *(Applausi)*.

di dittatura politica. Le buone norme inviterebbero a non intervenire con i decreti-legge soprattutto su materie sostanziali, materie ordinamentali, e soprattutto quella penale, e invece qui avete fatto di nuovo l'ennesimo errore.

decreto. La necessità, poi, non c'è nemmeno sotto un profilo di costituzionalità. Ricordiamo - come hanno fatto più volte i colleghi che sono già intervenuti - che il Presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di problematicità sull'impianto delle sanzioni, e non sull'impianto della norma. Si è discusso dell'entità della sanzione amministrativa. Oggi, inoltre, non solo non vi è questo tipo di urgenza giuridica e fattuale, ma non vi è nemmeno l'urgenza politica di provvedervi. di provvedervi. Il nostro Paese sta affrontando uno dei momenti più terribili della sua storia. Ci sono imprese che rischiano di chiudere; quasi il 30 per cento delle piccole imprese artigiane - per citare soltanto uno dei vari dati - pare non possa nemmeno più riaprire. Ci sono prospettive di disoccupazione che potranno dare anche degli indicatori molto preoccupanti. Ci sono dei dazi che pagheremo pesantemente nel futuro; un futuro che sarà veramente gravato da un debito pubblico che diventerà insopportabile, salvo che questo Governo non si ravveda e con fermezza decida l'utilizzo delle risorse eventuali che possono uscire dal *recovery fund* e che devono essere destinate alle aziende, perché l'ossatura di questo Stato sono le aziende, le imprese.

con quella insuperabile dottrina che da tempo purtroppo per certi versi inquina il vostro modo di pensare, non tenete conto di quello che viene detto dai cittadini. Credete di essere voi i depositari dell'intelligenza, i depositari delle grandi soluzioni

oggi una irragionevole ossessione, perché la vostra è un'ossessione: come avevate l'ossessione di Berlusconi, ora avete l'ossessione di voler cancellare tutto quello che è stato fatto dal ministro Salvini. ministro Salvini. La vera necessità, quindi, è per voi politica e strumentale di utilizzare e andare a distruggere quello che è stato fatto. I decreti Salvini funzionavano:

Vediamo i dati. A luglio di quest'anno sono arrivate 7.063 persone sulle nostre coste, contro le 1.088 dei tempi del ministro Salvini;

che la protezione speciale era stata introdotta con i cosiddetti decreti Salvini in modo da limitarla a serissimi casi, consentendo quindi ad alcuni soggetti di poter restare nel nostro Paese con un permesso. ci troviamo con dei permessi che sembrano richiamare quelli della protezione umanitaria; quella protezione umanitaria diventata labile, sbrindellata, molto ampia e generica.

se era previsto nel caso in cui la calamità riguardava eventi contingenti ed eccezionali, ora si tratta solo di eventi gravi. Che cos'è una calamità grave? La siccità è una calamita grave? È da considerarsi una calamità o una situazione che si è consolidata e che ormai è nella natura di un territorio? Non vogliamo che questi termini vengano utilizzati al fine di interpretare la norma più estensivamente e che ciò si traduca in permessi di lavoro.

capirlo bene. I cittadini sappiano che non sono ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione al diritto e al rispetto della sua vita privata familiare. Colleghi, cosa significa questo?

Sotto il profilo strettamente giudiziario vi erano delle possibilità di intervenire. Lo sappiamo. La Cassazione è ormai intasata di ricorsi in materia di immigrazione. Si è creato un meccanismo che lascia dei termini ampi e in questo modo un soggetto è libero di circolare sul nostro territorio finché non venga determinata la sua sorte in base a un ricorso giudiziale: questa è una problematica.

decreti Salvini sono stati votati, appoggiati e portati avanti da chi ora è fondante nella maggioranza con il Partito Democratico: il MoVimento 5 Stelle. corta. La memoria sarà corta, ma tutti ricordiamo - e ciò è ancora più imbarazzante - il Presidente del Consiglio che, se anche fa il Conte due, nel Conte uno

programma elettorale - non parlo del programma poi sottoscritto con la Lega, ma del vostro - c'era scritto «*stop al business dell'immigrazione»,* a firma Di Maio, capo politico Di Maio.

voi vergogna e non attaccare chi ha avuto il coraggio di venire dall'altra parte per difendere il Paese. Dovreste farlo anche voi; alzarvi da lì, venire qui, tirare fuori un pelo di dignità e non votare questa schifezza. Questo dovreste fare. Probabilmente però, come l'ex ministro Toninelli, avete sbattuto la testa e non ricordate più niente. Abbiamo visto anche lui scordarsi totalmente quello che ha firmato e cosa ha votato per quanto riguarda la questione dello *stop* agli sbarchi, i famosi porti chiusi,

decreti Salvini. Cercherò di farlo nel modo più semplice possibile, al fine che sia comprensibile veramente a tutti. Uno: anche la collega Stefani ha prima parlato di protezione umanitaria. la protezione umanitaria, anche nella questione delle ridistribuzioni, è stata un grande problema, perché la riconoscevamo solamente noi e, quando parlavamo di persone che avevano la protezione umanitaria, per gli altri Stati erano clandestini, essa non veniva riconosciuta. Tutti noi sappiamo che è una grande sanatoria, quella che piace tanto al Partito Democratico, e che ora il MoVimento 5 Stelle vuole mettere in campo. Una sanatoria che, però, cosa fa? Rende più insicuro il nostro territorio.

grazie a questo atteggiamento sull'immigrazione di una parte della sinistra, e ora pienamente anche del MoVimento 5 Stelle, trova braccia da rubare agli *hub*, ai centri dove si trovano gli immigrati, per metterli a spacciare sui territori. Siete complici di tutto questo *(Applausi)*; che non ve ne rendiate conto è la cosa grave, che non vi rendiate conto che state dando delle persone - alle quali non possiamo promettere un futuro migliore - in mano alla criminalità organizzata.

venivano mandati direttamente a Bologna. C'è un rischio sanitario. Questo non vuol dire, come piacerebbe a voi, che quando la Lega parla di rischio sanitario intende che gli immigrati portano malattie strane. Non è questo.

semplice: meno partono, meno muoiono; basterebbe guardare i dati. È quasi imbarazzante trovarsi qui a dovere spiegare a persone elette dai cittadini - che li dovrebbero rappresentare - una tale Dobbiamo aiutarli nel loro Paese? Sì. Non possiamo aiutarli da soli? Sì. Dobbiamo aiutarli insieme all'Europa? Sì. Ma questo lo dovete spiegare a chi con noi ha governato, e quando Matteo Salvini metteva in campo tutti i provvedimenti insieme a loro - lo avete scordato - per bloccare gli sbarchi, chiedeva ai Ministri 5 Stelle di aiutarlo sul fronte dei rimpatri, di aiutarlo a parlare con gli altri Stati, ma se ne fregavano, perché la vera questione è che la sinistra, come il MoVimento 5 Stelle, usa questo come baluardo, come bandierina, ma non gli importa niente né degli italiani, né di chi scappa realmente da una guerra. *(Applausi)*.

se difendiamo i nostri confini, difendiamo l'Europa; se non li difendiamo, mettiamo a rischio non solamente noi, ma tutta l'Europa. C'è un rischio terrorismo grandissimo, lo vogliamo negare? Vogliamo dire che siamo razzisti se diciamo questo?

in Europa, passando per il nostro Paese, che forse dovrebbe chiedere scusa perché non controlla i suoi confini. Dovrebbe imporre all'Europa di aiutarci e chiedere scusa per questo decreto-legge che sta votando ora in quest'Aula.

di emendamenti che parlavano di categorie chiuse, che hanno subito danni fino al 90 per cento nelle loro attività, se non di più,

un po' di mancette per mantenere, magari, le cooperative amiche; a voi non importa delle persone che vengono qua. Parlate tanto e vi riempite la bocca della questione della discriminazione per orientamento sessuale.

prima di procedere alla votazione, le chiedo la verifica del numero legale. Da questo momento siamo in fase di votazione, quindi procediamo all'appoggio da parte di dodici

di lavorare. Questo non è un modo di interpretare il ruolo di parlamentare. Il parlamentare deve finalizzare tutto ciò che fa alla realizzazione del suo compito.

C'è un problema sulla tribuna a sinistra: non c'è la connessione. A posto? No.

Grazie

le modifiche presentate dal Governo ai decreti sicurezza oggi in discussione sono l'emblema di una maggioranza in cui la sinistra ormai ha condizionato l'intero indirizzo politico e in cui il MoVimento 5 Stelle ha dimostrato di essere una bandiera che sventola a seconda del vento che soffia da destra o da sinistra. Prima di entrare nel merito della discussione, vorrei partire da due punti cardine della mia riflessione. Il primo punto è l'immigrazione, un tema molto importante per l'umanità, è parte del DNA dell'uomo e nessuno potrà mai fermarla. La politica ha il compito di gestirla e regolamentarla perché essa porti benessere alle persone che la vivono

che rappresentano persone e storie di vita; senza i numeri, le discussioni politiche corrono il rischio di fermarsi a percezioni emotive, dimenticando la politica reale.

né tanto meno possiamo negare gli oltre 20.000 morti in mare. Non possiamo nascondere gli elevati costi dello Stato per il sistema di accoglienza che, prima dei decreti-legge sicurezza Salvini, superavano i 4 miliardi di euro annui e che hanno illuso e abbandonato al loro destino centinaia di migliaia di giovani, in larga parte africani,

secondo il *global slavery index*, in Italia ci siano oltre 145.000 persone in condizioni prossime alla schiavitù; e subito penso a quei migranti, e non solo, perché oggi anche gli italiani corrono questo rischio. rischio. Vittime del caporalato e della tratta della prostituzione. Molti sono attratti nel nostro Paese con l'illusione di una vita migliore per i troppi segnali sbagliati di una pessima politica migratoria della sinistra. hanno saputo rispondere tempestivamente ai continui sbarchi sulle coste del Mediterraneo e hanno dato un segnale chiaro a tutti i Paesi di provenienza. Il sistema di protezione internazionale non è un canale di immigrazione economica, ma una via di arrivo di carattere emergenziale che genera lo *status* provvisorio di richiedente asilo, a partire da una domanda di asilo. Una politica seria deve distinguere l'immigrazione economica dal diritto d'asilo e differenziare i canali di ingresso per garantire protezione a chi ne ha davvero bisogno nell'attesa che possano cessare i conflitti nel Paese di origine e per assicurare che chi arriva in Italia possa vivere una vita dignitosa dal punto di vista economico. La sinistra, prima con i Governi delle scorse legislature e ora con il Governo Conte *bis*, vuole snaturare il sistema di protezione internazionale con ulteriori forme di protezione appositamente generiche e con la trasformazione della protezione umanitaria in permesso di lavoro, anziché impegnarsi sul fronte della politica estera per stipulare accordi con i Paesi di provenienza di applicare la legge che disciplina l'immigrazione regolare in Italia, quindi attraverso una possibile estensione del decreto quote per l'immigrazione fondata sul lavoro, che è immigrazione di qualità. Questo Governo vorrebbe fare del Mediterraneo, il *tunnel* della morte, il canale principale di arrivo nel nostro Paese dall'Africa. Ritengo profondamente ingiusto che si preferisca continuare a regalare false speranze a milioni di giovani africani, che rischieranno la vita nel mar Mediterraneo per un futuro totalmente incerto, anziché trattare con i Paesi africani per raggiungere condizioni che consentano davvero di trasformare l'immigrazione in una potenziale richiesta per il Paese. Sono i numeri a dirlo, cari colleghi: 6 milioni di immigrati irregolari in Italia producono il 9 per cento del PIL del Paese. È questa la strada su cui il nostro Paese deve lavorare per favorire i canali legali e sicuri, non quelli fondati sulle sanzioni, sulle sanatorie degli immigrati clandestini e sulle stabilizzazioni dei richiedenti asilo, che troppo spesso abusano dello strumento della domanda di asilo per eludere le norme sull'immigrazione che la politica non sa e non vuole applicare o aggiornare. Le regole non esistono per punire qualcuno, ma per il bene della comunità; la politica ha la responsabilità del bene comune, della salute e della sicurezza del popolo. I cosiddetti decreti Salvini, approvati dalla Lega, centrodestra e Movimento 5 Stelle avevano posto regole severe per scongiurare ulteriori morti in mare, per fermare gli sbarchi di migranti economici e portare il sistema di protezione internazionale alla sua funzione originaria. Oggi, cari colleghi, il vento che soffia da sinistra, la bandiera del Movimento 5 Stelle sventola dalla parte dei trafficanti di esseri umani, degli scafisti, delle cooperative del *business* di accoglienza della mano d'opera a basso costo, dalla parte di un sistema di protezione internazionale utilizzato per eludere le norme vigenti in materia di concessione di permesso di soggiorno e di lavoro.

Cari colleghi, stiamo riscrivendo la storia. Sì, l'antica storia infelice contro la dignità umana e io non voglio essere complice. Il lavoro è una cosa seria ed importante, perché esso consente di sostenere l'elevato costo della vita nel nostro Paese. Per tale ragione servirebbero accordi internazionali, per promuovere canali legali, fondati su incontro tra domanda e offerta di un vero lavoro, che consenta un'esistenza libera e dignitosa. La Lega auspica un'immigrazione fondata sul lavoro perché porta benessere e stabilità all'immigrato stesso e ricchezza al nostro Queste modifiche trasformeranno l'immigrazione in una causa di povertà e di emarginazione sociale. Queste modifiche lanceranno un messaggio molto pericoloso al di là del Mediterraneo, che l'Africa pagherà con migliaia di illusioni e di vite spezzate, che l'Italia stessa pagherà in termini di sicurezza e di spesa pubblica, soprattutto in un momento così difficile per il Paese. Cari colleghi, anziché approvare queste modifiche strumentali, finalizzate a riportare il nostro Paese alla pessima politica migratoria messa in atto per buona parte della scorsa legislatura, vi chiedo di ritirare questo decreto-legge, madre di una pessima politica migratoria non degna di un Paese civile, concentrandosi su tre punti che considero fondamentali: promozione dell'immigrazione fondata sul lavoro, quale condizione necessaria per un'esistenza libera e dignitosa degli immigrati in Italia e contrasto all'immigrazione clandestina; una politica estera che possa trovare accordi su cooperazione economica, rimpatri assistiti e ingresso regolare con i Paesi di principale provenienza, in connessione con le esigenze del nostro mercato del lavoro; infine, un sistema di asilo che anziché essere il principale canale di immigrazione senza alcuna...

possa davvero accogliere chi scappa da situazioni di conflitti o da persecuzioni reali, anche attraverso il canale umanitario.

è passato sommariamente per la fretta, per mandare avanti le cose, e non sono stati presi in considerazione punti molto importanti.

d'Azione in Commissione bilancio, e depositati anche nella Commissione di merito. Li leggo. Con specifico riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 2, in merito al trasferimento presso le strutture di sistema di accoglienza dei richiedenti, a seguito delle attività preliminari di assistenza, e alla lettera *c)* del medesimo comma, che afferma la necessità che i centri governativi ordinari e i centri straordinari siano caratterizzati da adeguati *standard* igienico-sanitari, precisando altresì quali siano i servizi che devono essere assicurati all'interno dei predetti centri, diversi sono i rilievi critici, che pare il caso di sollevare, alla quantificazione degli oneri presente nella relazione tecnica. Da un lato, non vengono esplicitati i criteri, che fissano al 7 per cento la stima dei maggiori costi relativi ai nuovi servizi di insegnamento della lingua italiana, di orientamento al territorio e di assistenza psicologica riconosciuti dalla disposizione in questione - tutto gratis, signori miei - d'altro canto, per definire la platea dei potenziali beneficiari, ai fini della quantificazione dei costi della misura, sono stati utilizzati come parametro i dati del 2019, determinando una cifra di 83.226 ospiti giornalieri medi, che appare decisamente sottostimata in considerazione delle serie storiche precedenti, del fatto che i dati del 2019-2020 scontano gli effetti delle politiche restrittive contenute proprio nei decreti che si intende modificare in senso estensivo con il provvedimento in esame determineranno con assoluta certezza un effetto incentivante del fenomeno. Basti solo considerare il tema dei ricongiungimenti familiari. Infatti, non appare chiaro come il maggior onere di 12,8 milioni di euro derivanti dalle presenti disposizioni possa essere coperto dagli stanziamenti presenti a bilancio, i quali non dovrebbero presentare risorse libere, anche in considerazione del fatto che il recente decreto-legge ristori *bis* e il decreto-legge ristori *quater* prevedono una riduzione proprio delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari di di 170 milioni di euro per l'anno 2020, quindi in completa contraddizione. A conferma di quanto sopra espresso, si evidenzia altresì che lo stesso Governo, nel disegno di legge di bilancio 2021, ha previsto un incremento di 100 milioni di euro annui delle risorse stanziate sul capitolo Fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo e degli interventi connessi, ivi compresi quelli attuati in adesione ai programmi e ai progetti dell'Unione europea in regime di cofinanziamento, confermando implicitamente che le disposizioni contenute nel presente provvedimento, a dispetto della presenza della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, sono assolutamente idonee a determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

senso. Le riprese parlano chiaro e le ho viste più volte anch'io. Voi però votate tutto, vi tappate il naso e votate qualsiasi cosa, pur di andare avanti con questo scempio. Sentitevi davvero complici. Siete complici del traffico di essere umani e delle morti in mare. Sentitevi complici!

siamo a fine anno, in piena pandemia mondiale

e pensate agli stranieri. Questa è la differenza, nel DNA, tra noi e voi!

che si mette al timone di un'imbarcazione non idonea ad affrontare il mare per la rotta che intraprende, sapendo che andrà incontro a delle difficoltà, ma avendo pronto il telefono satellitare per chiamare amici compiacenti e dir loro: aiutatemi a portare la merce e compiere l'ultima tratta (chiaramente per merce si intendono gli esseri umani). Si parte dalle coste settentrionali dell'Africa con il chiaro intento di commettere due crimini: traffico di essere umani, da una parte, e immigrazione clandestina dall'altra. Non vedo proprio come le convenzioni sul diritto del mare e della navigazione possano giustificare tutto questo. Mi permetto di dire che la questione non è nemmeno questa, in quanto il punto è politico. L'Africa ha circa 1.300 milioni di abitanti. Noi qui non stiamo parlando di aiutare un numero determinato o determinabile di cittadini che fuggono da un Paese in difficoltà per una guerra o qualche altro evento calamitoso; stiamo parlando di accogliere un numero potenzialmente indefinito di persone

l'identità di un popolo esiste e va protetta perché fa parte del patto sociale e della sicurezza che lega lo Stato ai cittadini. La sicurezza va garantita. In nome di presunti ideali o interessi economici, come molti miei colleghi della Lega hanno sottolineato in questi giorni, non può tollerarsi l'accoglienza indiscriminata, che non è accoglienza, ma, come ha sottolineato la senatrice Pucciarelli a inizio seduta, si traduce nell'ammucchiare esseri umani, contando di poter utilizzare i soldi pubblici per foraggiare una macchina di sfruttamento.

Fa specie che gli antirazzisti, gli antifascisti e i contrari a tutto siano i primi a incoraggiare l'immigrazione per poter avere manodopera a basso costo. Ridicoli!

Se i Padri costituenti, che pure venivano dell'esperienza della spagnola poco dopo la Prima guerra mondiale, non hanno previsto uno stato di emergenza per epidemia, forse un motivo c'è. L'unico stato di emergenza previsto dalla Costituzione con un procedimento particolare è quello in caso di guerra, che dev'essere dichiarata dalle Camere e poi dal Presidente della Repubblica,

Ecco un monito che mi venne fatto da un esponente locale della sinistra tanti anni fa, quando ero militante della Lega, a un gazebo:

Grazie è difficile parlare di cose che sono di un'evidenza scontata, soprattutto sapendo che chi ascolta non ascolta o è sordo o non vuole ascoltare. È del tutto evidente infatti che questo è un provvedimento che non ha né capo, né coda e sta dentro una logica che non è quella dei fatti, ma quella del provvedimento manifesto, che però - come dicevano benissimo i colleghi che mi hanno preceduto - in questo caso entra nel merito di alcune vicende che attengono alla convivenza civile e all'ordinamento dello Stato. Rispetto a tutto questo, colleghi, confesso di avere una certa difficoltà, perché non è possibile spiegare

Quando e se il mare lo consentirà, in Italia arriverà un'infinità di persone, senza alcun tipo di regolamentazione;

avete inserito nel provvedimento il motivo della discriminazione per l'orientamento sessuale; allora vedrete che ci sarà un proliferare di distinguo sul proprio orientamento sessuale. E come verificherete se la dichiarazione risponderà al vero o se sarà resa solo per avere la possibilità di essere ospitati? Come lo verificherete? Avrete soggetti soggetti che si presteranno a questo scopo? Avrete modo di verificare questa dichiarazione, come quella di provenire da Paesi in guerra, dove sono negate le libertà civili? rispetto a tutto questo, resta veramente difficile poterne anche solo parlare. Il problema sono le dimensioni del fenomeno, com'è stato osservato. Le nostre carceri sono per occupate da cittadini extracomunitari, gran parte dei quali, peraltro, è in carcere in quanto coinvolta nel traffico di stupefacenti. Come ha spiegato benissimo prima di me il collega Malan, i reati di violenza sulle donne sono compiuti per la maggior parte da cittadini extracomunitari. È inutile che scrollate la testa, come il cagnolino che una volta stava dietro la macchina (ricordate?). È inutile che scrollate la testa: è la realtà dei fatti. *(Applausi)*. Ho difficoltà anche solo a parlarne; infatti mi fermo qui

Oggi, 18 dicembre, l'Italia non sa che cosa potrà e dovrà fare il giorno di Natale. Anche qui è inutile che scrollate la testa come il cagnolino, perché noi forse consideriamo questo tema scontato, ne stiamo parlando da giorni e non se ne può più, ma fuori da qui la gente normale

l'Italia è ostaggio delle vostre beghe interne. Ieri avete tentato di fare una riunione, gli amici di Italia Viva hanno posto le loro condizioni e avete deciso Il Natale è ostaggio delle vostre beghe interne. Non so se avete contezza delle dimensioni della vostra inadeguatezza, perché questa è la realtà dei fatti; è inutile che continuiamo a girarci intorno. Non è la maggioranza, che non esiste, a essere ostaggio di Renzi. No, è l'Italia a essere ostaggio di Renzi, è il Natale a essere ostaggio di Renzi, malgrado Renzi.

che poi si è rivelato nella tempistica assolutamente perfetto. Ho auspicato di poter consentire ai nostri pescatori di passare il Natale insieme ai loro familiari

- ohibò! - a beneficio di telecamere, con Casalino in avanscoperta, addirittura con la geolocalizzazione. Benissimo, bravi, carini. Allora giocate con i cittadini italiani, che non devono sapere cosa possono fare a Natale, però il *Premier*, invece di risolvere le beghe e di stare seduto a Palazzo Chigi per tentare di risolvere i problemi, prende l'aeroplanino e va a rendere onore al generale Haftar, che i turchi hanno trattato da quel che merita. I turchi infatti gli hanno detto: "O liberi le mie motovedette, o in quattro giorni me le vengo a prendere"; e lui si è affrettato a liberare le motovedette dei turchi. Noi siamo andati invece a pagare prezzo, a pagare pegno. Abbiamo riconosciuto un'importanza istituzionale a un povero generalino da quattro soldi e l'abbiamo fatto a beneficio di telecamera, come se non bastasse. Vergogna, vergogna! Dopo 107 giorni. Vergogna! Non so più quante volte ve lo dovrei dire "vergogna". E allora stessero a casa!

perché, da un lato, vedo che un provvedimento che la maggioranza definisce così importante non ha mai visto, durante tutta la discussione - peraltro scarsa e scarna - in Commissione, la presenza del ministro Lamorgese. Lamorgese. Eppure, tecnicamente fa capo al suo Ministero. Abbiamo avuto la compagnia del vice ministro Mauri, che ho seguito anche durante i lavori della Camera,

Nel merito del provvedimento, voglio ricordare forse l'unica cosa che è venuta fuori dalla scarsa discussione in Commissione, cioè il fatto che il provvedimento in esame

- alla faccia degli appelli alla lettera del Presidente della Repubblica, che peraltro aveva fatto richiami ben diversi,

un'urgenza che di fatto, però, non c'è, perché, se è tanto urgente da andare ad agire su due momenti indicati dal Presidente della Repubblica nell'agosto 2019, evidentemente c'è qualche problema.

fuori nella discussione era se all'interno di quei barchini o barconi ci fossero o meno potenziali terroristi che utilizzassero questi canali, questi corridoi del mare e questi traffici umani

ha chiesto chi stabilisce che in quelle imbarcazioni che hanno accolto e salvato persone, naufraghi e profughi ci siano gli estremi per configurare un pericolo per il nostro Paese. Questa frase era nella dichiarazione sulla pregiudiziale pregiudiziale proposta anche dal Gruppo Misto, proprio in merito al fatto che tecnicamente non ci doveva essere pericolo all'interno di quei barconi *(Applausi)*, cosa che è stata smentita chiaramente. Credo che la maggioranza dovrebbe farsi un sano esame di coscienza, perché evidentemente l'inadeguatezza dell'azione e delle persone che agiscono in questo settore è ormai evidente. D'altro canto, è stato riferito anche da un membro della maggioranza - mi riferisco in particolare

«il vuoto pneumatico è esattamente il vuoto lasciato dalla vostra politica, il vuoto in cui l'illegalità ha prosperato. Per non parlare delle vergognose e disumane condizioni in cui chi dice di avere a cuore gli immigrati li ha costretti a vivere come bestie in gabbia». Questa era la senatrice Maiorino in merito a...

dell'ingresso legale nel nostro Paese. Devo dare atto alla relatrice, senatrice Valente, che nel suo intervento ha sostenuto la necessità di integrazione delle norme che si vanno ad approvare oggi e che vedranno il mio voto contrario. Devo apprezzare il suo intervento, anche se credo che bisogna tutti calibrare una nuova figura di parlamentare, perché negli ultimi tempi non abbiamo più uno scontro di visioni ideologico di idee,

anche la modalità di partecipazione al dibattito parlamentare ha un suo significato di pregnanza democratica. Nel 2008-2011, con l'ultimo Governo Berlusconi, non ho mai verificato la possibilità di porre la questione di fiducia prima della discussione generale: non si riteneva possibile. Nelle ultime due legislature abbiamo assistito anche a questo, compreso l'attuale provvedimento. Non c'è una Non c'è una regola scritta, ma la regola è che non si può prescindere dal confronto, se in esso si crede e se si ritiene che la nostra funzione non sia quella di affermare le idee del proprio gruppo,

come se ci fosse la possibilità che la funzione giurisdizionale sia svolta secondo le proprie idee politiche. È la negazione del diritto. Lo Stato di diritto è posto a fondamento della distribuzione del nuovo aiuto che l'Europa darà ai Paesi che hanno lo Stato di diritto, che significa che la funzione giurisdizionale non può mai essere succube o condizionata dalle proprie idee politiche. Se fosse così, sarebbe la fine del mondo. Nel momento in cui cioè un giudice, che svolge la funzione giurisdizionale, prescinde da questa verità, verità, sta alterando il rapporto istituzionale tra legislativo e giudiziario. Ciò è gravissimo.

allora a non rendervi conto che parlare di immigrazione significa definire anzitutto qual è il sistema che garantisce l'accesso legale al nostro Paese? Bossi-Fini non lo è: non funziona, va corretta e riscritta, perché dobbiamo tener conto oggi di una nuova situazione dei flussi migratori,

allora riequilibrare non attraverso bacchette magiche, ma attraverso la realizzazione di un'idea, discutendo come realizzarla.

con gli investimenti fatti nel centro dell'Africa e in Nigeria e con la realizzazione in Libia della famosa autostrada. autostrada. Bisognava creare lì infatti necessità di occupazione e possibilità di crescita per ridurre la forza del flusso migratorio verso il nostro Paese, la porta dell'Europa.

perché, al di là di della reale possibilità di accoglimento, non può esserci un ingresso legale. Non è questione di dare aiuto; l'aiuto si dà sul posto, collaborando perché ci sia un'iniziativa anche europea, oltre che dell'Italia, affinché si realizzino lì le condizioni minime di esistenza. Nello stesso tempo, dobbiamo realizzare un rapporto a livello europeo. La distribuzione nel nostro Paese ne presuppone una anche tra gli Stati europei

che altro non è che una correzione, perché volete fare finta che sia aperta. Badate, questa legge darà soltanto un'illusoria

che la nostra Costituzione pretende da ciascuno di noi, perché la funzione parlamentare sia svolta non nell'interesse di un partito o personale, ma in quello generale del Paese.

confesso di provare personalmente non poco disagio nel vedere il Parlamento impegnato su questo tema in un periodo nel quale la contingenza e la realtà suggerirebbero, invece, di concentrare ogni risorsa, ogni singolo sforzo, per aiutare il Paese a gettare le basi per una ripresa economica e sociale che dovrà essere importante e soprattutto ben strutturata. Ritengo necessario preventivamente sgomberare ogni dubbio da un concetto che qualcuno ha tentato di far maldestramente passare: da questo lato dell'emiciclo non siedono donne e uomini insensibili, non siedono mostri indifferenti al dolore o alle difficoltà; da questo lato, siedono semplicemente donne e uomini che mettono la sicurezza dell'Italia e dei cittadini italiani sempre e comunque al primo posto. «L'obiettivo del MoVimento 5 Stelle è quello di arrivare a sbarchi zero entro i prossimi cinque anni. L'immigrazione è il più grande fallimento dei partiti: hanno firmato accordi suicidi che hanno trasformato l'Italia nel campo profughi d'Europa e hanno foraggiato il *business* della criminalità organizzata. Quelle appena citate non sono mie parole. Era con frasi di questo tenore che veniva accompagnato, nel 2017, il programma immigrazione di uno dei partiti della maggioranza: frasi ben rappresentative di un concetto ripreso in maniera più analitica dal punto 8 del programma elettorale del 2018 di quello stesso movimento politico. Appare chiaro quale fosse la linea da seguire in tema di migrazione e, a onor del vero, va riconosciuto che, nei mesi successivi alle elezioni politiche, era stata tradotta, infatti, con la nascita dei decreti-legge sicurezza, fortemente voluti dall'allora ministro dell'interno Salvini e dalle forze politiche che supportavano quel Governo. La condivisione sul tema sussisteva ed è provata dalle numerose dichiarazioni audio, video e *social* o a mezzo stampa rilasciate da alcune delle personalità che più si adoperarono per quel progetto normativo, volte a esprimere una dura contrarietà nei confronti dell'accoglienza indiscriminata, che veniva etichettata come qualcosa da non dover mai più rivedere nel nostro Paese. Ci fu chi, forte di un ruolo da *leader* politico, in quel periodo richiamò all'ordine i suoi colleghi, tuonando che il MoVimento 5 Stelle era *pro* decreto sicurezza *(Applausi)*:«se c'è qualche membro della maggioranza a disagio sul decreto sicurezza, si deve ricordare che fa parte di una maggioranza che quel decreto lo ha votato, di un Governo che lo sta applicando, che lo sosteniamo e che chi prende parte, in questo momento, a questa *boutade*, prende parte a una *boutade* politica, per far sentire un po' di sinistra chi con la sinistra non ha più nulla a che fare». la stessa persona che nella scorsa legislatura, in tempi quindi non sospetti, non aveva avuto titubanze nel definire le ONG i *taxi* del Mediterraneo «chi dice che è inopportuno attaccarle fa finta di non vedere il *business* dell'immigrazione». Si tratta di quelle stesse ONG che oggi, con il provvedimento in esame, vedono alleggerite non poco le possibili sanzioni nelle quali potrebbero incorrere, nel caso di un eventuale illecito. Vi è poi chi, proprio negli ultimi giorni, ci ha dimostrato di non avere assolutamente più memoria di quel periodo, ma che all'epoca, in un'ospitata televisiva, difendeva così, con fierezza e fermezza, la paternità e la bontà del proprio operato: «Nel

la Lega non faceva niente. (...) Io sono responsabile della sicurezza della navigazione, fino all'attracco dell'imbarcazione al porto. Lui» cioè Salvini «è responsabile dopo, per la sicurezza dello sbarco e l'ordine pubblico. Se questi due elementi e queste due politiche non si integravano, non ci sarebbe stato questo 90 per cento in meno. Quindi, iniziamo a dire che è grazie al buon lavoro di due forze politiche, chiare e coerenti, che si portano a casa i risultati». In questa intervista il collega faceva riferimento a due forze politiche chiare e coerenti. Oggi però, a distanza di due anni, la storia ci racconta che solo una di queste due forze politiche è rimasta tale: la Lega. signor Presidente, è pacifico che non c'è nulla di illegale o di sbagliato nelle parole che ho sopra citato, anzi, tutt'altro: sono parole che condividevo allora e condivido oggi, parole condivise dalla stragrande maggioranza dei cittadini italiani, parole che elogiavano i decreti sicurezza semplicemente perché erano davvero provvedimenti che, indipendentemente da ogni retropensiero e colore politico, hanno reso l'Italia un Paese migliore e più sicuro dove vivere.

Era quella due anni or sono, quando il mio Gruppo di riferimento era un altro, ed è rimasta la medesima oggi, che sono parte del Gruppo Lega. Questo perché, su alcuni temi delicati, importanti e imprescindibili non può variare il giudizio solo in base al vento che soffia in un determinato momento politico. PRESIDENTE. Non dovremmo mai dimenticare che tutti noi siamo qui in rappresentanza dei cittadini italiani, che oggi ci chiedono supporto, prospettive e futuro, non di impiegare il nostro tempo e le nostre risorse per distruggere provvedimenti

Senatore Romeo ho visto il suo gesto di impazienza. Sto dando a tutti un minuto in più, ma vi prego di attenervi

vorrei preliminarmente sgombrare il campo da due obiezioni al decreto-legge in esame, che, da un lato, ne contestano i caratteri di urgenza e, dall'altro, lo accusano di essere mosso da spirito di rivalsa. Che in materia di immigrazione ci siano differenti impostazioni politiche e culturali tra le forze di Governo e di opposizione è fuor di dubbio, ma questo non dovrebbe portare a contrapposizioni ideologiche, poiché quello dell'immigrazione è un tema serio e complesso, che va affrontato di conseguenza. Che cosa si prefiggevano i due decreti sicurezza voluti dall'ex ministro Salvini? Direttamente, contrastare gli sbarchi di immigrati attraverso un controllo rigoroso dei porti, favorire il rimpatrio degli immigrati irregolari e contrastare il traffico di esseri umani. Indirettamente, avviare l'*iter* di modifica degli accordi contenuti e pretendere una distribuzione più equa dei migranti all'interno dell'area UE. Non voglio in questa sede soffermarmi sulle profonde lacerazioni sociali e culturali prodottesi in Italia a causa di una certa arroganza negli attuali respingimenti, né sul conseguente isolamento del nostro Paese nel contesto europeo. Voglio ricordare soltanto il dibattito interno al MoVimento 5 Stelle, fatto di perplessità e contrarietà ai provvedimenti in questione. Erano provvedimenti su cui però c'erano patti, il famoso contratto di governo. Ricordo i dibattiti laceranti

però stato un sacrificio inutile, perché, solo un mese dopo, ottenuto il risultato, l'ex ministro Salvini ha stracciato quel contratto di governo, provocando la crisi. Se l'intento dei due decreti era quello di impedire gli sbarchi e regolarizzare l'immigrazione, essi hanno fallito completamente l'obiettivo. Gli sbarchi dei clandestini e le morti in mare, pur contenuti nei numeri rispetto al passato, sono una piaga ancora viva nella nostra coscienza, nostra coscienza, mentre i rimpatri promessi non sono pervenuti. Al contrario, abbiamo assistito allo smantellamento del sistema dell'accoglienza e dell'integrazione. Non che non ci fossero in questo settore criticità e necessità di interventi migliorativi, ma l'enfasi - questa sì, ideologica - contro il cosiddetto *business* dell'accoglienza o le crociate contro le ONG hanno finito per buttare via, insieme all'acqua sporca, anche il bambino. Queste esperienze professionali, cresciute negli anni, che garantivano il passaggio dalla prima accoglienza a un percorso di integrazione sociale e lavorativo sono state frustrate. L'eliminazione della protezione umanitaria ha fatto sì che i richiedenti asilo, che in precedenza avrebbero avuto accesso a una forma di protezione, vale a dire a un permesso di soggiorno indispensabile per un percorso di integrazione, siano andati ad ampliare il bacino dei migranti irregolari. È quello che ha riconosciuto anche questo pomeriggio il senatore Malan, seppur con intenti diversi. Credo sia nata da qui una profonda riflessione, anche all'interno del MoVimento 5 Stelle, che ha portato al provvedimento attuale. sotto gli occhi di tutti che è stato snaturato il sistema ordinario e i centri di assistenza straordinaria gestiti dalle prefetture trasformati in contenitori dormitorio, dove i richiedenti asilo attendono l'esito della propria domanda di protezione internazionale: un percorso di tempo vuoto, che può durare un anno o anche più, in cui gli immigrati sono esclusi da percorsi di inclusione e lavorativi. asilo e rifugiati (SPRAR), riduzione dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) a una sorta di *bed and breakfast* contenitori, ridimensionamento delle figure professionali votate all'integrazione taglio delle ore lavorative di psicologi, mediatori linguistici e assistenti sociali hanno prodotto un esercito di immigrati invisibili, senza documenti e pronti a essere sfruttati. Con questo decreto immigrazione e protezione internazionale, invece, il Governo si propone, in un quadro di rinnovata concordia con i *partner* europei - che, paradossalmente, devo dire che nasce anche a causa della pandemia di sanare alcune evidenti criticità che sono fatti e non ideologie. Che si dovesse ridimensionare e rimediare a questo arretramento sociale e culturale ce lo dicono dunque i fatti. Con il decreto-legge su immigrazione e protezione internazionale al nostro esame si ripristinano i livelli della protezione umanitaria per i migranti che arrivano in Italia da Paesi considerati pericolosi, dove sono in corso guerre o persecuzioni, e si reintroduce il sistema di accoglienza e integrazione (SAI), un modello che tende a ricalcare quello degli SPRAR, reintroducendo la possibilità per i richiedenti asilo di accedere ai percorsi della seconda accoglienza, in un'ottica inclusiva e richiamando il precedente modello virtuoso di accoglienza. Sono premesse importanti, cari colleghi, ma non ancora sufficienti. Sarà necessario definire nel dettaglio i nuovi capitolati di gara: costi e servizi da erogare nei centri di accoglienza straordinaria e in quelli governativi. Solo rivedendo questi capitolati in maniera sostanziale sarà possibile portare i piccoli gestori e le relative professionalità a occuparsi dell'accoglienza diffusa. Il fenomeno delle migrazioni, però, non può essere gestito solo da decreti-legge, ma dev'essere accompagnato da una lungimirante politica internazionale. L'Italia, Paese che occupa il centro del Mediterraneo, non può rimanere spettatore inerte di fronte a quel che sta accadendo in Africa, nel medio e vicino Oriente. Ci illuderemmo, se pensassimo di gestire il fenomeno con misure esclusivamente interne. Occorre una più incisiva politica estera, capace di trasformare le nostre missioni internazionali da contingenti di interposizione volti ad assicurare la stabilità dei conflitti o l'addestramento delle forze dell'ordine locali onde prevenirli e contenerli in azioni di più ampio respiro. Senza l'impulso italiano, l'Unione europea continuerà a girare le spalle a questa fondamentale area del mondo, trascurando le politiche euromediterranee che tante aspettative avevano suscitato tra le due sponde del Mediterraneo. Altre forze stanno colmando l'assenza non solo nostra, ma dell'Europa: la Cina e la sua crescente influenza politica ed economica nel continente africano; la Turchia con il suo sogno neo-ottomano; la Russia, sul versante mediorientale; l'Arabia Saudita, con il sogno del grande califfato; Israele, col suo disegno di completamento dello Stato sionista con l'annessione progressiva dell'intera Palestina. Tutto ciò sta producendo nuovi venti di guerra nell'area, certamente non ininfluenti rispetto alla ripresa dei nuovi e più consistenti flussi migratori, di cui l'Italia sarà la prima a subire le conseguenze per la sua posizione geografica. non solo pensare, ma realizzare quanto prima un'agenzia europea dell'immigrazione con sedi operative in Africa per la migliore gestione del fenomeno, per quanto riguarda sia i corridoi umanitari, sia la politica dei rimpatri. a politiche attive dell'immigrazione, attraverso l'aumento dei contributi per la cooperazione allo sviluppo, anche tutelando i nostri imprenditori che mantengono rapporti commerciali con l'Africa e che possono creare occasioni di interscambio e crescita. Servono

mentre l'Italia è in ginocchio, mentre centinaia di migliaia di imprenditori sono disperati, mentre 5 milioni e mezzo di italiani sono precipitati sotto la soglia di povertà e le file per un pasto caldo si allungano a dismisura, il Governo e questa maggioranza artificiale e claudicante non trovano di meglio che occuparsi di immigrazione. E di occuparsene non per porre fronte E di occuparsene non per porre fronte all'aumento preoccupante degli sbarchi, passati dai circa 10.000 dello scorso anno agli oltre 30.000 di quest'anno, con gravissime conseguenze non solo di ordine pubblico e di sicurezza o di maggiori oneri per la finanza pubblica (alla faccia del vostro articolo 15 sull'invarianza finanziaria di questo decreto), ma anche e soprattutto di ordine con i molti focolai di contagio che in giro per l'Italia i migranti, gli unici che possono muoversi liberamente e fare tutto ciò che gli pare, hanno provocato in questi mesi (vedi Terzigno, Treviso, Fiuggi, Bolzano, eccetera). *(**Applausi)*. No, anzi. Voi al contrario vi preoccupate di aprire ancora di più le porte a tutti i disperati del mondo e tra loro, inevitabilmente, anche agli avventurieri e ai male intenzionati. Con questo decreto-legge voi accendete un radiofaro potentissimo

signor Presidente. Con questo decreto-legge voi accendete un radiofaro potentissimo verso l'Africa intera e tutto il Terzo mondo, per dire a tutti: venite quanti più potete, l'Italia è pronta ad accogliervi a braccia aperte, senza alcun limite. Questo voi state dicendo con questo decreto-legge. *(Applausi)*. Non solo chi fugge dalla guerra, come è giusto, ma che rappresenta solo il 5 per cento del totale; no, proprio tutti. Questo non è il decreto sicurezza, come voi falsamente lo avete definito; questo è il decreto invasione. Con queste norme potrà davvero entrare e rimanere in Italia chiunque la voglia. Basterà invocare una qualunque calamità, anche di modesta gravità, di cui ovviamente il mondo è pieno: un'estate troppo secca, un'inondazione, un raccolto andato a male o persino che nel proprio Paese non ci si può curare bene come in Italia. Questo prevedete. Oppure basterà lamentare anche il più piccolo torto subito in Patria, la più piccola discriminazione (vera o molto più spesso presunta) (vera o molto più spesso presunta) per il più disparato dei motivi. Avete persino inserito l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Basterà dichiararsi omosessuale, come in verità già avviene in molti tribunali, purtroppo, e non ci sarà più bisogno di dimostrarlo con questo provvedimento. Sarà, infatti, sufficiente, per la vostra aberrante logica, l'identità di genere, questa fumosa espressione che, com'è noto, è uno stato d'animo interiore, transeunte, soggettivo, indimostrato, indimostrabile e non verificabile. Basterà, ad esempio, presentarsi con i tacchi a spillo e con il rossetto per gli uomini o con un taglio di capelli maschile per le donne e il gioco sarà fatto. Oppure, ancora, avete previsto, non solo la necessità di curarsi da gravi patologie, come già avviene, ma addirittura da una qualsiasi malattia psicofisica. Basterà allegare un po' di depressione, patologia che non si può certo negare a chi chissà quali traversie avrà da raccontare, vere o presunte chi potrà mai dirlo, e il gioco sarà fatto: dentro un altro.

Cosa vuol dire? Non si capisce. Basterà, forse, lamentare il rischio di perdere la fidanzata o anche solo un amico. Ma vi rendete conto di cosa state facendo, cari colleghi? Lo chiedo soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che oggi voteranno in massa per cancellare anche quel poco di buono che avevano fatto. Anche voi avete abbracciato l'ideologia immigrazionista della sinistra. Capisco che Parigi val bene una messa, ma voi state innescando una bomba sociale di proporzioni inaudite. State richiamando in Italia centinaia di migliaia, milioni di migranti, destinati a competere per la sopravvivenza con i milioni di italiani al di sotto della soglia di povertà. E questo nel pieno della crisi economica più grave dell'ultimo secolo, con gli stranieri che scavalcano regolarmente gli italiani in tutte le graduatorie: dalla casa, alla scuola, ai servizi sociali. Stranieri ai quali è consentito persino l'accesso all'assistenza legale gratuita a spese dello Stato per fare ricorso avverso i decreti di espulsione fino in Cassazione; anzi,

se non bastasse, avete respinto la proposta di Fratelli d'Italia di fissare la soglia che ricordo essere la pensione minima che spetta agli italiani. Noi abbiamo chiesto di fissare questa soglia come indennità riconosciuta ad ogni migrante. Ma voi avete detto di no. Voi ai migranti riconoscete 1200 euro al mese Chissà perché: forse per alimentare il *business* dell'assistenza in mano a chi sappiamo bene? Cari colleghi della sinistra, questa è la verità. Gli affari dei vostri amici valgono un'invasione ai danni degli italiani per voi. E affinché sia del tutto chiaro che nessuno deve mettere ostacoli all'invasione, avete praticamente azzerato le multe a carico delle navi delle ONG che violano il divieto di ingresso nelle nostre acque territoriali, in modo che possano riprendere a pieno regime il loro ruolo ancillare a favore degli scafisti, raccogliendo in mezzo al mare il dolente carico di umanità alla deriva, laddove questi criminali, mercanti di vite umane, sanno di doverla lasciare, affinché poi le navi delle ONG possano raccoglierla e portarla a destinazione. Non capite che non basterà un'intera flotta per raccogliere tutti e che i naufraghi e i morti in mezzo al mare, anziché diminuire,

di Fratelli d'Italia avevamo avvertito, inascoltati, l'unico modo era e resta il blocco navale: solo impedendo le partenze si eviteranno le morti in mezzo al Mediterraneo.

caso, scusate, se lo ha fatto Prodi nel 1998 nei confronti dell'Albania, perché non possiamo farlo noi oggi nei confronti della Libia? Questo nessuno me lo spiega. Basterebbe la volontà di farlo, volontà che il Governo non ha, come dimostra la vicenda dei nostri pescatori, lasciati per oltre 100 giorni nelle mani di un signore della guerra che li ha sequestrati con un atto di pirateria e di fronte al quale il Governo è andato ieri a inginocchiarsi per ottenere di riportarli a casa. Questo è il Governo che voi offrite agli italiani alla vigilia del Natale, ma io vi chiedo di fare un regalo agli italiani: toglietevi di mezzo. non ho voluto interrompere il senatore Balboni, che stava concludendo il suo intervento, che abbiamo potuto ascoltare peraltro con interesse, ma non lascerò proseguire la seduta se non state seduti ai vostri posti. Ognuno rimanga seduto. Ho l'elenco di chi si è distinto per occupazione dell'emiciclo

rappresentanti del Governo, finalmente stiamo per realizzare - almeno in parte - uno degli obiettivi che la maggioranza si era posta quando ha dato vita al governo Conte-*bis*. Com'è noto, è stato uno dei motivi per cui Liberi e Uguali ha accettato di entrare nella maggioranza e sostenere il Governo. Con il provvedimento in discussione, pertanto, poniamo finalmente rimedio ai gravi errori che l'Italia ha commesso con i decreti "insicurezza" e con la pretesa di farsi scudo in Europa, non con la forza delle argomentazioni e della politica, ma sulle spalle dei naufraghi, sospendendo la cultura giuridica del nostro Paese, ripudiando la sua storia, rinnegando la sua umanità. Il Presidente della Repubblica fece delle osservazioni su quei decreti, che inviò con con una ben nota lettera al Governo e al Parlamento, soprattutto in relazione agli obblighi internazionali che il nostro Paese deve sempre onorare ed è un bene che questo provvedimento

ringrazio, Presidente, spero che mi faccia recuperare questo tempo. dicevo - si illuda però di risolvere con un decreto il complesso tema dell'immigrazione. Non lo facevano i decreti Salvini, non lo fa questo decreto per certi aspetti fin troppo timido. Serve un lavoro paziente, bisogna, a mio avviso, concentrare i propri sforzi su alcuni temi essenziali. Il primo è la revisione del Regolamento di Dublino, di cui tutti conosciamo l'importanza. Il secondo riguarda certamente il *memorandum* con la Libia, una vergogna che non posso omettere di ricordare e che penso che vada cancellato. Il terzo è la ripresa e l'aggiornamento costante dei decreti flussi. Il quarto è il superamento definitivo dell'impostazione della legge Bossi-Fini. Il quinto, non meno importante, è una nuova e più moderna legge sulla cittadinanza. Con questo testo facciamo passi avanti importantissimi, che hanno richiesto un difficile lavoro di sintesi e i cui esiti non erano per nulla scontati. Non posso tuttavia non segnalare un punto sul quale avrei voluto una maggioranza più coraggiosa e più determinata. In questi lunghi e difficili mesi, le organizzazioni non governative hanno coraggiosamente supplito alla drammatica inazione delle istituzioni comunitarie e nazionali, e nazionali, uomini e donne che hanno messo le loro energie e finanche il loro corpo a disposizione di un principio che è alla base della nostra cultura giuridica e della nostra società, quello dell'umanità. Le vite vanno salvate sempre, tutte.

molte persone e sofferto per ciascuna di quelle scivolate dalle loro mani restando in acqua. Ricordo a tutti noi le parole di Gaspare Giarratano, armatore di Sciacca che ha avuto seri problemi per aver salvato naufraghi con il suo peschereccio, ma che mai si è pentito di averlo fatto.

Anch'io, senatore Candiani, sono stato a Lampedusa. Ho assistito, da Presidente del Senato, allo sbarco di 125 migranti sul molo Favaloro e vi sfido a guardare negli occhi donne, uomini e bambini tremanti che hanno subito violenze indicibili e visto i propri cari morire. Vi sfido a chiamarli invasori. Ho visto anche, dopo l'offerta di un tè caldo da parte di volontari, quello sguardo di paura trasformarsi in una luce di riconoscenza e di speranza, speranza di sopravvivenza. Per questo ritengo che il punto non sia rimodulare le cifre delle multe previste, ma onorare chi salva vite umane e tornare al principio e allo spirito della Costituzione e affermare nuovamente e sempre i valori fondamentali della nostra comunità.

finalmente voteremo questo provvedimento, nonostante le continue provocazioni di queste ore, e dimostreremo la volontà del Parlamento e del Paese di cancellare una pagina vergognosa, quella dei cosiddetti di cancellare la grande menzogna che cerca di scaricare sui migranti la rabbia giusta di chi non ha lavoro, le difficoltà di chi è precario, intermittente, partita IVA, artigiano, e combatte ogni giorno, specie in questo tempo di pandemia. Avete alimentato veleno, come le pazzesche teorie complottiste sullo scambio etnico, sull'immigrazionismo. Ma la realtà è un'altra ed è sotto gli occhi di tutti. La questione migratoria è un fatto epocale e non sarà fermata da nessun muro, perché le cause che la generano sono più forti dei muri, e sono guasti come guerre e calamità, guasti di un modello di sviluppo spesso predatorio di cui siamo responsabili e che l'Occidente ha imposto al resto del mondo. E va governata senza mai derogare allo Stato di diritto, alla nostra identità democratica. Noi oggi cancelliamo l'ignominia di decreti Salvini che hanno ostacolato il salvataggio di vite in mare, un atto sacro da sempre, da quando esiste la nostra civiltà, un atto virtuoso ed eroico secondo le leggi dell'uomo e il codice del mare. Avete criminalizzato il volontariato che salva vite, come le ONG, che con la loro azione meritoria hanno supplito ad un obbligo che spetta alle istituzioni. Criminalizzando chi accoglie, avete rovesciato i nostri valori e infangato l'onore dell'Italia, alimentando paura e xenofobia, mistificando e avvelenando lo spirito pubblico. Quei decreti-legge sono infatti il simbolo dell'inganno ai cittadini, in particolare i più deboli, messi gli uni contro gli altri in una falsa rappresentazione; e sono stati lo sfregio della Costituzione nei suoi valori più identitari, che sono stati messi in discussione. Chi impose a tutti i costi quei decreti-legge, facendone l'immagine nefasta della prima parte di questa legislatura, ha voluto chiamarli "decreti sicurezza", ma con la sicurezza non hanno mai avuto niente a che fare; anzi, hanno causato, all'opposto, caos e illegalità, perché la cancellazione della protezione umanitaria, e contestualmente lo smantellamento del sistema di accoglienza e della rete di integrazione incardinata sui Comuni, ha messo in una condizione di illegalità e di clandestinità, e dunque anche di pericolosità sociale, la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo, fuori da ogni controllo da un sistema di inserimento sociale che noi oggi, con questa legge, ricostruiamo. I cosiddetti decreti Salvini hanno ridotto migliaia di persone in manovalanza per il lavoro nero, per il caporalato, per la criminalità organizzata - altro che sicurezza innescando tante bombe sociali nei territori e nelle città, specie nelle zone più complicate dove c'è più frustrazione e dove è più difficile È per questo che i primi strenui oppositori sono stati i sindaci, che hanno cercato di scongiurarne l'approvazione, e poi immediatamente ne hanno chiesto la cancellazione. Questo da subito è stato anche il nostro impegno, l'impegno del Partito Democratico, prima dall'opposizione e poi come condizione per la formazione del nuovo Governo, come netta e necessaria discontinuità da quello precedente. Rigettando i cosiddetti decreti Salvini, noi respingiamo e cancelliamo il tentativo pericoloso di criminalizzare la povertà trattandola come un fatto di ordine pubblico e non invece come questione sociale; come se vivere in condizioni di disagio fosse una colpa da punire e non invece una stortura, un mal funzionamento dell'intera società. Questa legge segna finalmente un'estensione dei diritti con l'introduzione dell'istituto della protezione speciale, che amplierà, rafforzandola, la norma precedente, quella delle protezione umanitaria, che era stata colpita dai decreti Salvini. Questa norma ripristina nella sua interezza uno dei cardini della nostra Costituzione, il diritto d'asilo per chi vede negate in patria le libertà fondamentali e lo rafforza tornando a legarlo a quanto discende dagli obblighi e dai trattati internazionali, come più volte, con voce netta, ha richiamato il presidente Mattarella. Noi abbiamo il dovere politico e morale di cancellare leggi sbagliate, di non essere indifferenti e immobili di fronte al dramma delle stragi che si susseguono nel Mediterraneo. Questa legge può essere la base di una nuova politica migratoria, che rafforzi il ruolo e la credibilità dell'Italia nel Mediterraneo, che ottenga una politica migratoria europea, archiviando il Regolamento di Dublino, rilanciando la cooperazione internazionale con l'Africa, riattivando i corridoi umanitari e i cosiddetti decreti flussi per l'emigrazione economica. il modo più efficace per stroncare i trafficanti che prosperano sull'illegalità e per questo va finalmente cancellata la cosiddetta legge Bossi-Fini che non solo è sbagliata nell'ideologia, ma non ha mai funzionato, tanto è vero il Governo del centro destra è ricorso a due maxi sanatorie negli anni scorsi e quella legge costringe ancora nella irregolarità migliaia di lavoratori stranieri, che potrebbero concorrere al nostro sviluppo e al nostro sistema previdenziale e pensionistico. Signor Presidente, serve rilanciare le ragioni dell'Italia e dell'Unione europea, che è nata proprio dal rifiuto del nazionalismo, del filo spinato, contro genocidi e campi di concentramento, contro oppressioni e discriminazioni razziali. Non possiamo essere inermi di fronte alla perdita di vite in mare e alla violazione dei diritti dei migranti in Libia, che sono i nostri stessi diritti. Sono stragi che saranno ricordate come una colpa imperdonabile e di fronte alle quali non si potrà dire: "non sapevamo", perché noi sappiamo. L'Italia nel 2013, con l'operazione Mare Nostrum, seppe dimostrare la propria forza e la propria grandezza morale e politica, salvando migliaia di naufraghi. Oggi, cancellando di fatto i decreti Salvini, riacquista onore e reputazione. Oggi torniamo a lavorare per costruire sicurezza nell'unico modo possibile e duraturo attraverso inclusione, integrazione, riconoscimento reciproco di diritti e doveri inderogabili dopo questo, servirà finalmente una legge sulla cittadinanza che permetta...

Questa è l'Italia: potenza politica ed economica perché amata, rispettata e riconosciuta nel mondo per la forza dei suoi diritti e dei suoi valori, che voi avete tentato di negare e di infangare e che noi oggi in quest'Aula riaffermiamo.

onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, trattiamo di un decreto-legge sicurezza a distanza di poco più di un anno dal varo di un precedente decreto-legge sicurezza. la cosa che fa specie è che questo Governo, in un momento emergenziale, in cui i problemi sicuramente non mancano, ha ritenuto urgente modificare un provvedimento che una parte importante di questa maggioranza, un anno fa, aveva partecipato a realizzare. Vi dirò di più. Circola sui siti e sui *social* il video di un'intervista di un tal ministro Toninelli. Pensavo, come la maggior parte degli italiani, che la battaglia contro l'immigrazione clandestina fosse stata un cavallo di battaglia di Salvini e della Lega. No, Toninelli dice che è stato un suo successo. Dice che se è avvenuto il blocco dell'immigrazione clandestina è stato grazie al Governo del cambiamento, grazie al MoVimento 5 Stelle. ha un problema di coerenza, perché quando approverete questo decreto-legge, e ci sarà, invece, l'immigrazione incontrollata, dovrà dire che il merito è del Governo della restaurazione, quella che il MoVimento 5 Stelle ha fatto con il Partito Democratico per mantenere la poltrona. Amici del rinnovamento, amici del cambiamento, se questa è la coerenza, se questo è il nuovo, ridateci il vecchio; almeno era coerente con se stesso e non si sarebbe mai contraddetto in maniera così evidente come state facendo

strumentale un richiamo del Presidente della Repubblica che, in occasione del varo del primo decreto-legge sicurezza, per non rimandarlo all'esame delle Camere, disse che forse era necessario rivederlo in due punti, esclusivamente la quantificazione della sanzione amministrativa e le cause di non punibilità. Ebbene, avete utilizzato questa raccomandazione del Presidente della Repubblica come un grimaldello per demolire quello che era stato realizzato. Avete reintrodotto la protezione umanitaria, la ristrutturazione del sistema di accoglienza in piccoli centri diffusi sul territorio, un ridimensionamento delle multe alle ONG e avete eliminato il provvedimento di sequestro. Colleghi, c'è una differenza fra il Paese che state creando voi e uno dei Paesi più civili, come la Germania. Vi faccio un esempio: in Italia, Carola Rackete, che ha forzato un blocco navale e ha speronato le nostre navi da guerra, abbiamo messo un tappeto rosso e l'abbiamo mandata a casa. *(Applausi)*. per il semplice fatto di aver partecipato a un corteo di protesta contro l'abbattimento di alberi è stata arrestata. Questa è la serietà di un Paese civile; ci sono le leggi e le leggi vanno rispettate. State creando le condizioni per fare di questo Paese l'Eldorado dell'immigrazione clandestina. Ci sono numerose criticità. Mancate di una visione strategica; avete ampliato le casistiche del permesso di soggiorno e avete soppresso il termine stabilito al 30 novembre per indicare le quote di flusso che l'Italia avrebbe potuto sostenere e supportare.

la povertà si è allargata da 5 milioni a 5,5 milioni, abbiamo perso 500.000 posti di lavoro, e l'anno prossimo ne perderemo 1 milione, vi preoccupate di garantire gli immigrati che vengono qui. non sempre perché scappano da guerre. Vedete, colleghi, un'altra cosa che mi fa specie è il richiamo all'articolo 10 della nostra Costituzione, cioè a quell'articolo che dice che chiunque scappa da una guerra e da una persecuzione ha diritto di essere sostenuto e di essere accolto. voi che portate avanti questa politica irrazionale sull'immigrazione, siate quelli che vogliono salvaguardare i diritti umani e noi siamo quelli che invece li vogliamo pregiudicare. Quasi che voi vogliate salvare i disperati in mare e noi invece li vogliamo annegare. *(Applausi)*. Noi siamo per salvare questi disperati, ma siamo per salvarli con una normativa che eviti di metterli nelle mani degli scafisti senza scrupolo, come voi state facendo. come voi state facendo. *(Applausi)*. Non è neanche il caso di paragonare questa migrazione alla migrazione italiana, iniziata nel 1860, che si è protratta fino al 1961. I nostri antenati sono entrati nei Paesi stranieri in punta di piedi, si sono adeguati, si sono integrati, hanno lavorato anche facendo lavori umili e degradanti. Questa gente viene in Italia e, dopo essere stata accolta, ci vuole imporre di rinunciare alle nostre tradizioni e alla nostra cultura! *(Applausi)*. Vuole eliminare il crocifisso dalle scuole, non ci vuole consentire di fare il presepe e questo non è un modo di fare accoglienza.

di una politica strategica, vogliamo incentivare l'immigrazione, ma quella buona, quella delle intelligenze e delle persone che vengono per integrarsi e per farlo devono innanzitutto riconoscere e accettare la nostra cultura, le nostre origini e la nostra tradizione; devono imparare la lingua italiana e la storia del nostro Paese. *(Applausi)*. Solo in questa maniera si potrà dire realizzata una effettiva integrazione, che non è quella che state praticando. Anche l'autorevolezza del nostro Paese nel contesto europeo è cambiata di molto

esultando quasi per un Accordo sottoscritto in quel di Malta, che avrebbe consentito la ridistribuzione degli immigrati su tutto il territorio europeo. la redistribuzione c'è stata, ma soltanto all'interno del nostro Paese, con oneri a carico dei Comuni e delle piccole realtà territoriali *(Applausi)*, alle quali sottraete risorse alle quali sottraete risorse e servizi, dando garanzie, che non hanno neanche gli italiani, agli extracomunitari. Voi pregiudicate i nostri connazionali e questa è una responsabilità che vi porterete dietro e della quale darete conto, prima o poi, al popolo italiano. In questi giorni sto rileggendo la biografia di Winston Churchill e all'interno di questa lettura ho trovato un episodio, che credo si presti molto al periodo che stiamo vivendo. Correva il 1940, era iniziata la seconda guerra mondiale, le cose non andavano bene per l'Inghilterra

"avete occupato per troppo tempo quelle poltrone, per quel poco che avete fatto per il Paese. È arrivato il momento che vi dimettiate". Sono convinto che, così come fece Chamberlain che accettò quell'invito, prima o poi il primo ministro Conte farà Voteremo no all'ennesima fiducia, su un provvedimento inutile, non necessario e assolutamente non conforme al diritto.

che il Paese affronterà, nel momento in cui c'è la crisi economica più pesante di sempre e le angosce degli italiani sono sulla loro esistenza, è lo *ius soli*. Complimenti! Questa è la capitolazione definitiva del MoVimento 5 Stelle tra le braccia del Partito Democratico. Siamo veramente alla farsa ed è incredibile perché, invece di chiedere conto a un Governo che ha delle responsabilità enormi nell'aver riattivato il *business* degli immigrati clandestini e degli scafisti, con il loro terribile carico di morti, voi oggi smantellate quelle stesse leggi che, fatte dalla Lega e da Matteo Salvini, Ministro dell'interno, hanno salvato vite umane impedendo gli imbarchi. Complimenti! Paradossalmente, arriviamo oggi a votare qui in Senato dopo che il processo a cui voi avete mandato Salvini a Catania ha cominciato a rivelare quella che è la matrice politica che ne sta alle spalle, con

questo provvedimento nasce da un tradimento, che è denominatore comune per il MoVimento 5 Stelle nel Governo Conte due: quello delle giravolte, degli impegni rimangiati e dei tradimenti. È successo per la TAV: vi siete rimangiati tutto. È successo per il gasdotto TAP: vi siete rimangiati tutto. È successo per la vicenda Ilva: vi siete rimangiati tutto. È successo per Alitalia: vi siete rimangiati tutto. È successo per Autostrade e per quel ponte Morandi che mi fa venire in mente il senatore Toninelli, di cui non ricordo nemmeno il nome. il superamento della regola del secondo mandato, di cui vi siete scordati anche il significato, e per il contrasto agli scafisti e all'immigrazione clandestina,

avere la faccia di presentarsi in Aula a smontare quello che loro stessi hanno approvato in Consiglio dei Ministri. *(Applausi)*. Dov'è il presidente del Consiglio Conte, che è il primo firmatario di questo disegno di legge "clandestini"? Dov'è il ministro Lamorgese? Dov'è Bonafede? sono Di Maio, Guerini, Speranza, Patuanelli e Gualtieri? Dove sono? Tutte poltrone vuote. Questo è il bell'esempio che date agli italiani. Complimenti!

Questo è quello che sta accadendo oggi qua dentro. C'è poi un altro tema, quello della sinistra che non si ricorda più che cos'è la sinistra e che, con la visione con la visione accecata dall'odio verso l'avversario politico, perde il senso della realtà fino ad andare a impostare politiche migratorie che avranno un solo fine,

costringere le persone al sussidio; costringere le persone a essere mantenute e, per gli italiani che non accettano questo regime, ad andarsene. Questo è quello che state facendo. Questa è la sinistra *radical chic* di cui dovete andare fieri, ma non potete scappare alle urne. Là dentro arriverà il responso. Approvate questa legge, approvatela contro gli italiani e gli italiani che porteremo al *referendum* per abrogare questa legge vi presenteranno il conto. Lo presenteranno a questa sinistra che inconsciamente odia tutto ciò che è identità italiana. Volete cancellare i decreti sicurezza contro Matteo Salvini?

State tornando a commettere gli stessi errori, quelli che ci avevano portato nelle piazze gli spacciatori; quelli che ci avevano riempito il Paese di delinquenti clandestini; quelli che hanno portato in Italia gente che poi abbiamo visto andare a fare gli attentati negli altri Paesi europei. State compiendo ancora gli stessi errori e non c'è dibattito qua dentro che riesca a farvelo capire, perché voi avete perso il contatto con la realtà. E l'unica cosa che vi interessa oggi è imporre visioni ideologiche, perdendo di vista che oggi l'Italia si trova nella peggiore crisi economica di sempre, come ho già ricordato. È lo stesso paradosso che vi ha impedito di capire quando, all'inizio della pandemia Covid, dicevamo di chiudere le frontiere. Vi dicevamo di chiudere le frontiere verso la Cina

Complimenti! È la stessa visione lucida che vi porta oggi a modificare questi decreti sicurezza e ad andare a fare i decreti per i clandestini. Complimenti! I numeri vi condannano, quelli pubblicati sui siti del Viminale, quelli che ci dicono che sono 33.000 quest'anno gli sbarcati e che erano 11.000 lo scorso anno. Questi sono i numeri che vi condannano.

accalcati, schiacciati, senza dignità, senza alcuna possibilità di veder rispettati quei diritti di cui poi vi lavate la bocca qua dentro. Ma nessuno di voi è andato a Lampedusa nessuno di voi è andato a Lampedusa a vedere qual era l'effetto del decreto che volete oggi approvare con la fiducia, una volta che gli immigrati sbarcano in Italia. Non ci siete andati perché avete paura a guardarvi allo specchio e a guardare la vostra realtà. Fermatevi, fate ancora in tempo. Non date ulteriore carne da macello agli scafisti. Vi troverete presto a rispondere di queste responsabilità e allora non basteranno i «non so», «non ricordo», «non c'ero e, se c'ero, non ho capito», «non c'ero e non mi ricordo», come lo smemorato Toninelli. Ma che tristezza quella della bugia detta per nascondere la propria incapacità di prendersi una responsabilità! E che tristezza quando questa responsabilità è quella che chiedono gli italiani di difendere il proprio Paese. E nel frattempo dove vanno gli scafisti? Dove li state nascondendo? Li state nascondendo nel cono d'ombra del Covid. Non c'è dibattito, non c'è informazione sulla stampa, non c'è nulla sulla cronaca. Ma sappiamo che i 30.000, una volta che sono stati liberati dalla quarantena, sono in giro per l'Italia con un foglio di carta in mano, dove si dice loro di tornare nel proprio Paese e quelli nel proprio Paese non ci tornano ed entrano in clandestinità. facendo, senatrice De Petris, ed è il contrario di quello che qualcuno ha detto qua dentro. Questo vuol dire mettere in clandestinità le persone e obbligarle poi a finire tra le braccia della malavita organizzata. State riempiendo un'altra volta le fila degli immigrati clandestini e della criminalità organizzata. Questa è un'altra responsabilità da cui non potrete fuggire. Non c'è dubbio, Presidente: voi oggi portate in approvazione questa modifica della norma dei decreti sicurezza per un odio ideologico.

oggi ci troviamo qua in Aula ad approvare un decreto trasformato in legge senza che ci sia stata nemmeno una discussione generale Non ha alcun valore andare a vedere i precedenti, perché l'unica cosa che dicono i precedenti è che oggi voi, MoVimento 5 Stelle, con il vostro ministro D'Incà, state utilizzando i peggiori metodi della Prima Repubblica, quelli che mettono il bavaglio all'opposizione, quelli che impongono la fiducia, quelli che impediscono qualsiasi dibattito anche alla maggioranza. *(Applausi)*. Non una parola abbiamo sentito dal MoVimento 5 Stelle oggi qui in Aula. Questo è l'imbarazzo che vi inchioda alle vostre responsabilità. Potrete tradire voi stessi, ma pagherete sempre il conto di aver tradito gli italiani. Prego i senatori Questori e gli assistenti parlamentari di procedere

Prego, senatrice Questore, rimuova al posto di indicare me.

Quando abbiamo finito con i cartelli, passiamo ai fischietti. Incarico lei di andare a trovarli. Finiamola con questi cartelli. Forza, senatrice Pergreffi, si costituisca. Con i cartelli abbiamo finito. Adesso non ricominciamo. Ascoltate: la mia intenzione è di non sospendere la seduta e di proseguire, sperando che una volta o l'altra Cristiano Militello ci noti, perché vedo che a "Striscia lo striscione" non ci siamo mai andati. Forse si doveva mettere qualche errore. Tanto alla fine poi vi stancate. Riprendete fiato, per cortesia.

i toni canori di questa parte della discussione possono e debbono essere soppressi. Colleghi, legittima è l'esternazione di un dissenso, ma, oltre un certo punto, stona.

con questo provvedimento, finalmente, vince la sicurezza, quella vera, e perde la paura, quella che serve solo alla propaganda elettorale. Come tanti altri, anche noi abbiamo contestato i decreti Salvini, dicendo che avrebbero peggiorato le problematiche connesse all'immigrazione. In particolare, con quei decreti ...

In particolare, con quei decreti-legge si chiusero gli SPRAR, quei piccoli centri di accoglienza dove tante persone lavoravano con successo per l'integrazione dei migranti e che fungevano anche da antenne per il controllo del territorio. Inoltre, con il fortissimo restringimento dei permessi umanitari, tante persone furono catapultate nell'invisibilità, facile preda della criminalità organizzata alla ricerca di forza lavoro a basso costo. Per non parlare delle norme sul salvataggio in mare, in contrasto con gli accordi internazionali; tanto che - com'è noto - il presidente Mattarella scrisse una lettera alle Camere per sollevare forti perplessità, sollecitando il Parlamento a modificare il provvedimento. Per fortuna, questa stagione si è chiusa, nonostante i patetici tentativi di ostruzionismo da parte di chi ha fatto della paura il proprio *business* elettorale.

tutto con particolare attenzione ai minori non accompagnati e alle persone più vulnerabili. Si lasciano alle spalle i grandi centri di accoglienza, tanto pericolosi per il fatto di tramutarsi in fonti di conflitto sociale - anche per via delle condizioni non sempre ottimali di quei luoghi si punta sui piccoli centri diffusi, che sono più semplici da gestire e diminuiscono i rischi di tensioni con il territorio, tornando a prevedere corsi di studio non solo per i rifugiati, ma anche per i richiedenti asilo, che invece erano tagliati fuori dai decreti sicurezza. Torna anche l'iscrizione all'anagrafe sanitaria dei richiedenti asilo, perché era semplicemente folle che vi fossero persone che non avevano diritto all'assistenza sanitaria. Siamo rientrati nel perimetro della Carta costituzionale, vietando il respingimento di persone in luoghi nei quali rischiano di essere sottoposte a tortura o ad altri trattamenti inumani e degradanti. Il permesso per motivi umanitari, per chi non ha i requisiti per ricevere lo *status* di rifugiato, è semplicemente una questione di civiltà. Inoltre, sappiamo che l'espulsione ha efficacia solo verso i Paesi di provenienza con cui l'Italia ha stretto accordi bilaterali. Su questo fronte anche il bilancio dell'ex Ministro dell'interno, nonostante i tanti annunci, è piuttosto carente. nonostante i tanti annunci, è piuttosto carente. L'unica via, quindi, è lavorare per l'integrazione di quelle persone, mettendole al riparo dalle mire delle organizzazioni criminali. Di buon senso è anche la norma che consente la conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro e anche qui nulla di particolarmente sconvolgente: siamo sulla scia di quanto fece un Governo di centrodestra con la legge che portava il nome di Umberto Bossi e Gianfranco Fini. L'attività di soccorso in mare viene liberata dal pesante giudizio negativo; vengono abolite le sanzioni assurde per chi salva le vite, mai applicate perché in evidente contrasto alle leggi internazionali del mare, come descritto perfettamente dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento nelle motivazioni della non convalida dell'arresto di Carola Rackete. L'aiuto in mare, il diritto-dovere di soccorso, viene ripristinato come atto costitutivo della nostra idea di società. Con questo provvedimento la violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali viene punita con una multa molto ridimensionata e, soprattutto, non potrà più essere applicata alle operazioni di soccorso. Positiva è anche la stretta nei confronti di attività criminali, con l'inasprimento del Daspo urbano per gli spacciatori, anche in assenza di una condanna definitiva; così come positivo è l'inasprimento delle norme per i soggetti coinvolti nelle risse, un intervento dedicato a Willy, il ragazzo di origine capoverdiana ucciso a calci e pugni da un gruppo di delinquenti alcuni mesi fa. Purtroppo la popolazione ha la sensazione che ai criminali non succeda mai nulla, che vengano arrestati e rilasciati il giorno dopo per continuare con lo spaccio, con l'occupazione in piazze cittadine e comportamenti intimidatori e aggressivi nei confronti dei passanti. Ne sappiamo qualcosa a Bolzano, dove siamo rimasti tutti indignati per l'aggressione verbale sessista a un assessore comunale da parte di un gruppo di migranti, cui è seguita una retata delle forze di polizia. Contro questi criminali si deve agire con fermezza e rigore. Non è accettabile che nella popolazione, per colpa di tali personaggi, si affermi l'idea dell'immigrazione come sinonimo di criminalità, perché i migranti sono soprattutto quelli che si prendono cura dei nostri anziani, lavorano nei nostri ristoranti, puliscono le nostre case e i nostri alberghi. Questi stranieri sono quelli che pagano anche i contributi e le imposte e, in un Paese dove purtroppo non si fanno più figli, il loro contributo è essenziale anche per il sistema pensionistico. Sfatiamo poi questo luogo comune: con una lettura attenta dei dati ci si rende conto che gli stranieri non commettono più reati degli italiani. Inoltre, se si entra nel merito dei reati commessi dagli stranieri, il 70 per cento è commesso da irregolari. È la riprova che, quando una persona è esclusa da qualsiasi possibilità, quando c'è il divieto di lavorare o di trovare forme legittime per il proprio sostentamento, la conseguenza diretta è la devianza sociale. Per concludere, Presidente, con questo provvedimento si è ristabilito un principio di umanità e civiltà che non dovrebbe mai mancare in un Paese con la storia e la maturità democratica dell'Italia. È l'inizio di un nuovo percorso, in cui mi auguro davvero che la questione smetta di essere un elemento della più becera propaganda e diventi un tema da affrontare con intelligenza e rispetto della sua complessità. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.

quello di oggi non è un voto contro, quello di oggi è un voto per: un voto per chi scappa da condizioni disumane alla ricerca di una vita dignitosa e di un futuro migliore, ma è anche un voto per il Paese, per i nostri interessi, per ripristinare di fatto sicurezza e legalità; quella sicurezza e quella legalità che nel fumo della propaganda degli anni scorsi erano invece state compromesse. La scommessa che abbiamo di fronte è di non farci travolgere dagli arrivi, ma al tempo stesso non lasciare che muoiano altri migranti in mare e non creare nuove sacche di irregolari; una partita che è molto più complessa degli *slogan* a cui c'eravamo dovuti abituare due anni fa nel corso della continua campagna elettorale a cui ci costringevate. Il ministro dell'interno Lamorgese, in appena un anno di lavoro, è riuscita a conseguire due risultati importanti: ha riportato la questione migratoria nella sua sede naturale, cioè la cornice europea, ed è riuscita a ridurre di dieci volte il numero di decessi in mare rispetto al suo predecessore, attraverso il superamento della logica dei porti chiusi; un risultato di rilievo, anche se resta ancora drammaticamente insufficiente dal momento che ogni vita persa è una perdita di troppo, ma è un risultato che auspicabilmente potremmo andare a migliorare proprio con questa legge. una legge che innanzitutto sana i rilievi sollevati sui decreti Salvini dal presidente Mattarella e dalla Corte costituzionale; quei rilievi che il Presidente aveva contestato al Governo e al Parlamento in merito alla cancellazione del diritto umanitario e al rispetto dei trattati internazionali,

sia con la confisca delle navi alle organizzazioni umanitarie. Con questo decreto, allora, l'Italia torna ad essere un Paese rispettoso del diritto europeo e internazionale. Il provvedimento sana pure i rilievi della Corte costituzionale, che aveva bocciato il passaggio che impediva agli stranieri richiedenti asilo di registrarsi all'anagrafe. Ecco che con le modifiche che andremo a votare ripristiniamo diritti e legalità: anche ammesso che l'intento dei decreti Salvini fosse quello di porre un argine all'illegalità, di certo essi non hanno raggiunto tale obiettivo; anzi, hanno creato ampie sacche di illegalità attraverso l'abolizione, nell'ottobre del 2018, della protezione umanitaria. Fino ad allora ne beneficiavano circa 20.000 immigrati all'anno e il decreto ha avuto l'effetto disastroso da un punto di vista pratico, tanto che chi era in attesa di un riconoscimento - e prima della legge lo avrebbe ottenuto con la scomparsa della protezione umanitaria si vedeva opporre un diniego, diventando clandestino a tutti gli effetti. Il risultato è stato creare almeno 37.000 nuovi irregolari in soli due anni, a cui si sono aggiunti tutti coloro che già precedentemente godevano di una protezione umanitaria, e cioè circa 39.000 persone, ai quali non è stata rinnovata. Quindi, oltre oltre 70.000 irregolari sono sostanzialmente frutto dei provvedimenti dell'allora ministro Salvini: persone invisibili, destinate a sparire nel nulla, perché i rimpatri nel frattempo non sono aumentati. Sono quindi soggetti di cui non abbiamo informazioni, con tutti i possibili pericoli che questo può comportare, come si è visto purtroppo recentemente nell'attentato terroristico a Nizza, il cui autore era risultato essere entrato in Europa dall'Italia. Ecco perché è cosa buona e giusta che si vada a reintrodurre la protezione umanitaria. È positivo per i diritti dei diretti interessati, che acquistano così identità, ma è ottimo anche per la sicurezza del Paese, che potrà così identificare e monitorare i migranti che sta accogliendo. Altrettanto positive sono le ulteriori modifiche che andiamo a prevedere con questa legge: prima fra tutte l'introduzione della SIA, il Sistema di integrazione e accoglienza, che ripristina sostanzialmente gli SPRAR, un'ottima rete di piccoli centri di accoglienza diffusi sul territorio che erano stati - anche questi - aboliti dai decreti Salvini. la questione migratoria è un fenomeno complesso, un fenomeno che attiene alla sfera dei diritti ma anche dei doveri; una complessità che non può trovare risposte semplici, banali. Per questo la modifica dei decreti sicurezza, frutto di un lungo lavoro di mediazione tra il Governo e le forze di maggioranza - lavoro per il quale mi sento di ringraziare sia il ministro Lamorgese che il sottosegretario Mauri - è un primo passo importante, a cui sarà necessario farne seguire altri. Innanzitutto serve urgentemente la riforma del Trattato di Dublino, cosicché tutti i Paesi europei possano partecipare al processo di accoglienza. Qui bisogna dire che, ancora una volta, non sarà facile conseguire questo risultato, dal momento che i Paesi di Visegrad, stretti amici di Lega e Fratelli d'Italia a livello europeo, sono tra i più duri oppositori alla revisione del Trattato stesso. E, quindi, è tutto da verificare che si riuscirà a modificarlo, e soprattutto a modificarlo in una versione che sia favorevole per l'Italia. Poi serve una riforma della legge sulla cittadinanza che consenta a migliaia di ragazzi e ragazze, nati e cresciuti nel nostro Paese, di essere riconosciuti a tutti gli effetti come cittadini italiani. Infine, bisogna investire sulle politiche per l'integrazione: integrazione nel mondo della scuola, del lavoro, nel sociale e nelle rappresentanze, perché è solo attraverso l'integrazione che i migranti possono dare il meglio di sé e si possono rivelare in tutta la loro potenzialità, come una risorsa preziosa per il Paese di accoglienza, oltre che per il singolo. Ne sono la prova quelle centinaia di migliaia di nostri connazionali che decine di anni fa furono essi stessi migranti alla ricerca di lavoro, in giro per l'Europa e per il mondo. Giusto qualche giorno fa proprio qui, nelle aule del Senato, abbiamo celebrato i sessantacinque anni degli Accordi bilaterali tra Italia e Germania per il reclutamento di lavoratori italiani; lavoratori che dal 1955 partirono come *gastarbeiter* per contribuire alla ricostruzione della Germania postbellica. Al nostro evento hanno partecipato dirigenti, professori universitari, giovani *manager*, sindaci, relatori che ci hanno raccontato la storia di quei nostri migranti, i loro genitori o nonni, nel corso dei decenni. La maggior parte sono storie di successo, proprio grazie all'integrazione raggiunta. Quelle esperienze ci insegnano, ancora oggi, alcune cose di grande attualità: in primo luogo, se si guarda all'immigrazione solo come a un pericolo e ci si rifiuta di adottare misure per l'integrazione, si possono generare problemi di lunga durata insuccessi scolastici, disoccupazione, marginalizzazione sociale dei giovani migranti, disagio, violenza ed eventualmente anche criminalità. Se invece, viceversa, si guarda all'immigrazione come a un'opportunità e si lavora per l'integrazione, allora si creano le basi per il successo professionale dei migranti e se ne ricavano ingenti benefici per l'intera società, in termini sia di crescita economica che di coesione sociale. Questa è esattamente la storia dei tanti nostri connazionali in Germania, ma anche in tanti altri Paesi dove i nostri connazionali si sono affermati brillantemente. io credo che questa storia, così caratterizzante per il nostro Paese - una storia di migranti che, nonostante le tante difficoltà, sono riusciti ad affermarsi con successo non vada dimenticata, e anzi ci serva oggi per capire quanto l'immigrazione possa essere una ricchezza non solo per sé, ma anche il per il Paese in cui si sceglie di vivere. vivere. Se è vero che gran parte dei risultati di chi emigra è frutto della forza di volontà dei singoli, è anche vero che parte della loro riuscita dipende dalle buone politiche di integrazione che sono state messe in atto dai rispettivi Paesi di accoglienza. Credo che sia utile che la nostra esperienza di Paese di emigrazione ci serva da faro per mettere in campo buone politiche per l'integrazione che, oltre a valorizzare le tante potenzialità dei nostri migranti, creino al contempo le migliori condizioni, anche sociali, per la crescita e lo sviluppo del Paese, esattamente come hanno contribuito a fare negli anni tantissimi nostri emigranti italiani in giro per il mondo. *(Applausi)*.

possibile che una persona di un altro pianeta, di un altro sistema della galassia, oggi venisse ad ascoltare quello di cui stiamo discutendo, penserebbe che veramente questa umanità, prendendoci per la generalità degli umani, è pazza e irresponsabile.

le famiglie sono divise e, ad oggi, non sanno se a Natale potranno raggiungere i propri parenti; mentre gli imprenditori tengono le aziende chiuse e stanno fallendo; mentre coloro che hanno avuto la certezza di poter aprire i locali e i ristoranti a Natale, e hanno già comprato le derrate alimentari, le devono buttare perché pare che

nel luogo dove gli italiani dovrebbero essere rappresentati, il problema più urgente oggi, con la malattia imperante, con i problemi di Natale che aumentano le difficoltà, è discutere

da metà di coloro che oggi sono nella maggioranza. Anzi, si tratta di più di metà di quelli che oggi sono nella maggioranza, i quali sono stati ben felici di prendersi dei meriti in quel caso e oggi, con un po' di imbarazzo - almeno spero devono prendersi i meriti del provvedimento opposto e contrario. La sinistra, che dà sempre, pervicacemente, antepone interessi ideologici al bene dell'Italia e al bene degli italiani, non ha questi problemi. e non ci vengano a dire che è nell'interesse di chi ha subito persecuzioni nel proprio Paese o fugge da una guerra. Non abbiamo mai negato a costoro il diritto di asilo. Non abbiamo mai negato il diritto di venire in Italia a chi veramente ha un motivo riconosciuto dalle leggi internazionali. Basta guardarsi in giro per capire che è una scusa flebile e bugiarda. Sanno tutti benissimo che già ora, in giro per le nostre città - bella accoglienza - c'è gente disperata in mano alla malavita o che gironzola, dorme dove capita, e non ha niente a che vedere con coloro ai quali è riconosciuto il diritto d'asilo. E siccome questo non bastava,

Non stiamo parlando di bloccare una mamma con un bambino che fugge dalla guerra: ci mancherebbe! Stiamo bloccando l'espulsione e consentendo

Qualcuno ha ricordato cosa è successo a colei che ha speronato la nave: in Germania l'hanno arrestata per molto meno. Per carità, c'erano delle multe? Quasi non ci sono più. Per carità, c'erano dei provvedimenti giudiziari? Non più. In una parola sola, il dato ideologico, sempre voluto dall'internazionale marxista, prima, e di sinistra, oggi è: aboliamo le frontiere. Non c'è identità nazionale; non importa dove sei nato, non importa che lingua parli, non importa che cultura hai o quale religione pratichi; non importa l'italiano o un'altra lingua, l'ho detto. Ma non importa nemmeno se rispetti le leggi fondamentali o no; dovunque tu sia, sappi che in Italia puoi venire. Se non è un diritto all'invasione questo, ditemi voi cos'è. Chi ci guadagna in tutto ciò? Gli scafisti *(Applausi)*, ma anche coloro che vivono sull'accoglienza. Non a caso abbiamo proposto che venisse equiparato il costo dell'immigrato clandestino alla pensione minima di 546 euro. No, per l'immigrato 1.200 euro; evidentemente i soldi non vanno in tasca ai poveri immigrati; finiscono al *business* dell'accoglienza, sul quale si stenta moltissimo Presidente, spezzo una lancia a favore degli immigrati veri, quelli non clandestini. Mi ha scritto un cittadino albanese, si chiama Jimmy, abita a Ragalna, a via Paternò - lo potete cercare - e mi ha detto che, benché abbia un lavoro,

gli hanno negato il rinnovo del permesso di soggiorno perché guadagna poco; quindi, c'è una persecuzione verso gli immigrati regolari per favorire quelli che sbarcano clandestinamente e che magari vanno a fare attentati in altre parti d'Italia. *(Applausi).* che, con l'avvicinarsi del Natale, tutti devono stare lontani, a casa, guai a salutare i parenti. È stato detto che 70.000 uomini delle Forze armate vigileranno. Possibile che non se ne trovino 7.000 per per controllare che non scappino dai centri di accoglienza coloro che vi sono e dovrebbero rimanere rinchiusi? *(Applausi).* Possibile che non si accolga la proposta di Fratelli d'Italia almeno di riconoscere economicamente gli straordinari ai militari, alle Forze dell'ordine che, poveretti, passeranno il Natale a impedire che si veda il fratello o la nonna,

Non mi piace generalizzare le responsabilità, perché nel PD c'è una componente ideologica,

paura che spetti agli italiani decidere se potranno mantenere o meno la poltrona. Capisco che questo non rechi vergogna

ed è a Capo di un altro Governo, che vuole abolire con eguale forza questi decreti-legge. C'è una persona, che si chiama presidente Conte, che dopo questa ennesima figuraccia dovrebbe avere il buon gusto di dimettersi. Conte, dimettiti! rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, prendo la parola per dichiarare il mio voto, quello delle colleghe e dei colleghi di LeU e di altri senatrici e senatori del Gruppo Misto. un voto favorevole alla fiducia chiesta dal Governo, un sì convinto. Oggi, finalmente, torna a risplendere la luce, dopo questo periodo buio che ci lasciamo alle spalle con i decreti Salvini, la cui unica sicurezza era quella della propaganda continua, che ha creato solo insicurezza, disparità, disprezzo e odio nei confronti degli ultimi e di chi, le ONG, si sono sostituite agli Stati, andando in mare e rispettando la legge del mare: salvare le vite umane. Nel corso del dibattito sono intervenuti nel merito del decreto-legge colleghe e colleghi del Gruppo Misto. Mi preme sottolineare qui l'impianto di queste norme. Signor Presidente, con il voto di oggi saniamo la ferita inferta al nostro Stato di diritto, alla nostra cultura giuridica liberale, perché consideriamo i soggetti a cui sono destinate queste norme degli esseri umani. Sono stati anni terribili, nei quali si sono messi i penultimi contro gli ultimi, donne e uomini che avevano un lavoro e un percorso di integrazione entravano d'improvviso nell'ombra, diventavano invisibili e chi aveva un documento di protezione umanitaria poteva perderlo, finendo nel circuito dell'illegalità, quindi espulso dal sistema di accoglienza. Irregolari da un giorno all'altro, senza diritti per renderli ricattabili, il capro espiatorio delle sofferenze e dell'abbandono delle nostre periferie. Siamo orgogliosi dell'impegno umanitario delle ONG della società civile. Non vogliamo le ONG per mare? L'Europa torni a schierare le flotte, come fece all'indomani della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, 368 morti. Noi non dimentichiamo l'*hangar* dell'aeroporto dell'isola siciliana, con tutte quelle bare. Tutti i potenti d'Europa dissero: mai più! «Provo vergogna e orrore», dichiarò il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che aggiunse: «è necessario rivedere le leggi anti-accoglienza». Sì, dovremmo prima o poi mettere mano alla madre di tutte le leggi antiimmigrati, la Bossi-Fini, una legge criminogena. *(Applausi)*. Il nostro Paese, all'indomani di quella strage, autorizzò l'operazione Mare nostrum, per evitare il ripetersi di altri tragici eventi nel Mediterraneo. Poi all'operazione Mare nostrum si sostituì quella a guida europea, Frontex, e poi via via, se prima eravamo in dieci, oggi sono rimaste solo le ONG. Altro che in combutta con gli scafisti! Nessuna ONG è sotto processo; altri lo sono oggi. *(Applausi)*. È importante che sia legge il fatto che non si possano applicare le misure di interdizione all'ingresso nelle acque territoriali alle navi che effettuano soccorso in mare nel rispetto delle norme del diritto e delle Convenzioni internazionali, il che significa che l'equipaggio che sta per effettuare un intervento di salvataggio lo deve comunicare al proprio Stato di bandiera e che la stessa cosa deve fare con il centro di coordinamento competente per il soccorso marino, di cui deve seguire le indicazioni. Certo, c'è ancora molto da fare a livello nazionale ed europeo sul fronte dell'integrazione e di una gestione dei flussi migratori all'insegna del diritto, della ragione e dell'umanità, ma siamo sulla strada giusta perché questo decreto chiude, speriamo per sempre, la stagione in cui si è criminalizzato l'immigrato e perché finalmente si affronta il fenomeno delle migrazioni con razionalità, nel rispetto dei principi della civiltà giuridica e del diritto internazionale. Migliaia di persone - donne e uomini con nomi e storie drammatiche - erano diventate improvvisamente invisibili, disprezzate e definite con una parola che dovrebbe essere cancellata: clandestini. *(Applausi)*. Ho ascoltato con attenzione i colleghi dell'opposizione

dell'interno Salvini che fine aveva fatto la promessa di allontanare dall'Italia il mezzo milione di irregolari? Quanti ne avete rimpatriati? È facile fare propaganda, giocare sulla paura della gente e sulla disperazione e mettere gli uni contro gli altri, ma così non si affrontano le questioni, le si amplificano solamente.

deputati, migliorando ulteriormente il testo), ha consegnato a Palazzo Chigi 4 permessi di soggiorno speciali: alla vedova di Thomas Daniel, la signora Cinzia, e ai tre colleghi di lavoro del giovane liberiano scampati alla morte. Thomas Daniel e Ciro Perrucci, napoletano, erano i due lavoratori edili morti a Napoli il 1° giugno scorso mentre realizzavano una palazzina abusiva. Thomas e Cinzia erano arrivati in Italia diciotto anni fa dalla Liberia e avevano il permesso di soggiorno per scopi umanitari. Poi, con i decreti Salvini, divennero sfruttati sfruttati e invisibili. Le crisi economiche e sociali, i cambiamenti climatici e le guerre spingono moltitudini di persone a spostarsi e a lasciare le loro comunità alla ricerca della sopravvivenza. È la storia dell'umanità, È la storia dell'umanità, che è sempre stata scandita dalle migrazioni fin dalle epoche preistoriche. E allora, piuttosto che fare propaganda, bisogna governare questi fenomeni: cambiare il regolamento di Dublino, aprire corridoi umanitari, impegnare l'Europa e approvare finalmente una legge sulla cittadinanza. Signor Presidente, aspettavamo da mesi la cancellazione dei decreti Salvini, da quando cioè è nato questo Governo, e oggi finalmente ci siamo. Lasciamo alle spalle la disumanità.

un sistema diffuso di tanti piccoli gruppi per limitare al massimo la conflittualità. Di fatto, c'è la reintroduzione della protezione umanitaria, anche se in questo decreto si chiama speciale. E, ancora, aver reso molti permessi di soggiorno convertibili in permessi di lavoro favorisce l'integrazione, l'integrazione, che è la nostra arma migliore. Mi avvio a concludere l'intervento. Conservo in me diverse immagini: le bare di Lampedusa, il ghetto di Rosarno, il corpicino senza vita di Alan Kurdi, il funerale di Thomas Daniel. Vorrei leggervi una frase, quella di Pam, una giovane vietnamita che ha lasciato sul telefonino alla sua mamma prima di soffocare nel *container*, trasportato da un TIR: «Mamma e papà, perdonatemi se il mio viaggio verso un Paese straniero finisce qui. Non respiro più. Sto morendo. Mamma mi dispiace tanto. Vi amo tanto». Sì, noi dobbiamo rispondere alle Pam, agli Alan e alle tante vittime innocenti della povertà. C'è bisogno di umanità, di far emergere dal sommerso e dal nero migliaia di uomini e donne sfruttati e sudditi. *(Applausi)*. Marginalizzarli vuol dire consegnarli al circuito criminale consentire loro di entrare nel circuito legale vuol dire stessi diritti e doveri degli altri. Colleghe si celebra la Giornata internazionale per i diritti dei migranti. Noi non porteremo mai pazienza se qualcuno morirà per colpa nostra. Il diritto a vivere e il diritto a sognare il futuro sono universali. Noi stiamo dalla parte delle persone. Noi, colleghe e colleghi, votiamo sì alla fiducia posta dal Governo.

subito il voto favorevole del Partito Democratico alla fiducia al Governo e al provvedimento un provvedimento importante che contiene anche norme rilevanti su altre questioni: penso per impedire l'ingresso in carcere di telefonia abusiva e quelle che danno più strumenti al Garante per tutelare non solo i detenuti, ma anche chi è istituzionalizzato nelle RSA. però chiaro che questo provvedimento contiene soprattutto misure per governare meglio, con giustizia e umanità, l'immigrazione, un fenomeno con cui tutte le società occidentali si confrontano e si dovranno confrontare per ragioni demografiche, sociali e di squilibri internazionali. Se è così, una parte importante della discussione fatta in questi giorni non ha senso. Se è così, il tema non è dividersi tra chi vuole aprire e chi vuole chiudere. Nessuno vuole aprire o aumentare l'immigrazione, come state dicendo, e nessuno è stato capace di chiudere, come state dicendo. Il tema non è chi vuole o chi non vuole il clandestino. Nessuno di noi vuole i clandestini. Il vero punto e la vera differenza è tra chi vuole agitare il problema e chi invece vuole governarlo. *(Applausi)*. voluto da tutta la maggioranza (e ringrazio il MoVimento 5 Stelle per aver onorato un impegno), cancella norme contenute in due decreti-legge che - diciamolo subito - non hanno prodotto nulla di buono, ma sono serviti per fare propaganda. Sono stati il manifesto di chi indica un nemico su cui scaricare paure e preoccupazioni. Nessun problema di criminalità, disordine, clandestinità è stato risolto, anzi; ce l'avete detto voi. Noi oggi interveniamo per cambiare provvedimenti che hanno cambiato in peggio e umiliato uomini e donne che già sono qui, già risiedevano in Italia, anche se venuti da altri Paesi. Si è chiusa una parte importante del sistema di accoglienza e di integrazione, abbandonando sul nostro territorio migliaia di persone che avevano diritto a restare. *(Applausi)*. Si sono tolti i permessi umanitari a persone integrate che, grazie a quei permessi, potevano lavorare e mantenere la famiglia.

la clandestinità, la precarietà, altro che rispettare chi ha davvero bisogno, chi lavora e vuole integrarsi! *(Applausi)*. Avete consegnato all'illegalità migliaia di persone. L'idea è che bisogna trattare male quelli che sono qui per evitare che altri siano invogliati a venire qui. Quelli che secondo alcuni di voi, come ho sentito in questa discussione, decidono di partire, attraversare il deserto, mettersi nelle mani di schiavisti o scafisti e rischiano di morire in mare fanno tutto questo perché vedono la televisione o perché il nostro Paese rispetta i principi di umanità. Non è così e lo sapete benissimo. Partono perché sono disperati e neanche quei rischi li possono fermare. Poi c'è l'altra parte, gli altri nemici da esporre alla rabbia degli italiani: le ONG, le organizzazioni che hanno

ma lo si racconta lo stesso, perché a qualcuno bisogna dare la colpa e mica si può darla alla fame, alle guerre o alle dittature. Serve un nemico più vicino, che ha l'unica colpa di salvare le vite di persone sgradite. Poi c'è la realtà: i decreti Salvini non sono serviti a risolvere neanche uno dei problemi qui elencati dall'opposizione. come dicevo prima, hanno reso più debole l'integrazione sul territorio e il controllo. Questi decreti non hanno reso gli italiani più sicuri. Non è che, se non si parla continuamente di immigrati tenuti in una nave, vuol dire che il problema dell'immigrazione non viene risolto, mentre invece, se si parla tutti i giorni di navi tenute al largo con gli immigrati, si sta risolvendo il problema dell'immigrazione. Gli auditi stessi e una parte di quest'Aula hanno descritto una situazione di degrado e di difficile integrazione; hanno parlato della stazione Termini e degli sbarchi aumentati. Ricordo che tutto ciò fino a ottobre è accaduto mentre erano in vigore i decreti Salvini, perché fino a ottobre erano in vigore i decreti Salvini. *(Applausi)*.

D'altra parte è molto complicato governare l'immigrazione e dovrebbe saperlo il centrodestra, perché chi oggi denuncia una situazione difficile è anche l'autore di tutte le norme che intervengono in materia di sanità e di di sanità e di immigrazione, dai decreti Salvini alla Bossi-Fini. Siete voi gli autori delle leggi in vigore. Non basta agitare i problemi; serve lavorare con l'Europa. Le dichiarazioni del presidente von der Leyen sul fatto che l'immigrazione è un problema europeo e non dei singoli

Vanno eseguiti i rimpatri, come ha fatto il ministro Lamorgese. Nei primi otto mesi del 2019 (credo ci fosse un altro Ministro) sono stati fatti 541 rimpatri al mese; negli altri quattro mesi, con questo Governo, sono stati fatti 651 rimpatri al mese, a testimonianza del fatto che non è sulla legalità la differenza tra noi, ma sull'umanità. *(Applausi)*. E siamo anche d'accordo sul fare entrare legalmente solo chi vuole lavorare. Ma oggi non è possibile entrare legalmente in questo Paese per un immigrato. non c'è sicurezza, se si viene meno ai principi di umanità. C'è sicurezza se questo fenomeno viene governato, non agitato e utilizzato per alimentare consenso sulla pelle delle persone. Noi cerchiamo di governarlo. Speriamo che anche voi e i cittadini capiate che il tema è questo: governare l'immigrazione, non agitarla. Agitandola, e con disumanità, si creano solo più problemi di quelli che si pretende di risolvere.

Noi ieri abbiamo applaudito, convintamente, alla liberazione dei nostri pescatori, che erano dei liberi lavoratori imprigionati ingiustamente e che non davano fastidio a nessuno. Ancora oggi, l'agenzia

dopo un processo in Italia per traffico di clandestini. Chiedo, in quest'Aula, al Governo se ciò è vero o non è vero. Non conosco questo giornale. Leggo le agenzie italiane. di uno scambio di prigionieri. Noi difendevamo lavoratori sequestrati. Questi, invece, erano scafisti condannati per tratta di persone e vengono messi, forse, sullo stesso piano. Questo decreto-legge si può riassumere in una frase: più lassismo, che comporta più partenze di clandestini dal Nord Africa, più viaggi e, senatore Ruotolo, più morti. Il numero dei morti, infatti, con il numero dei viaggi e con la politica del lassismo nei confronti dei trafficanti di persone. La vostra retorica non la accettiamo, perché è la vostra politica che ha moltiplicato le tragedie nel Mediterraneo. Lo voglio dire chiaramente: contrordine, compagni, come avrebbe detto Guareschi, perché quelli che si spacciano per i buoni, per definizione, sono i cattivi, che, con il loro lassismo, moltiplicano le tragedie. E noi, che saremmo i cattivi, siamo i buoni, che vogliono bloccare la tragedia delle morti nel Mediterraneo: è la nostra politica che lo può assicurare. Nel 2020, l'anno che sta per chiudersi, gli sbarchi saranno quasi 40.000; nel 2019, erano stati 10.000. Quei decreti, che voi volete abrogare con questo voto, erano, quindi, migliori di queste norme che adesso sono già in vigore. Voglio poi ribadire che noi, come Forza Italia, anche al Governo giallo verde, ma, nel merito di quei decreti, dicemmo che apprezzavamo una politica di fermezza nei confronti dei clandestini e del traffico di persone, perché era uno dei baluardi del programma politico unitario. Contestammo, Contestammo, in quel decreto, la mancanza di soldi e di risorse alle Forze di polizia. E dico qui al Governo: non avete ancora ricevuto il comparto sicurezza e difesa per rinnovare il contratto. Avete violato le leggi. Non li avete ricevuti al varo della manovra di bilancio. È inutile dare pacche sulle spalle al popolo in divisa, anche in questi giorni di emergenza. Date loro soldi e contratti, che avete negato finora a tutto il comparto sicurezza e difesa. quindi, non solo è una misura politica, ma è una misura ideologica e, come abbiamo discusso ieri in sede di questione pregiudiziale, è anche immotivata la necessità e urgenza. Il decreto-legge è pasticciato e confuso e tratta varie materie. Se volete fare un decreto-legge per necessità e urgenza, lo dico anche al vice ministro Misiani, vi do un suggerimento: guardate i prezzi di treni e aerei in questi giorni e le speculazioni per la gente che deve tornare a casa. Fate un decreto-legge per impedire la speculazione sui prezzi dei trasporti: lì c'è necessità e urgenza. La gente deve comprare il biglietto e non sa ancora quando, quando deciderete che cosa si deve fare.

dai bastioni di Malta, durante una bella conferenza stampa annunciò l'accordo per la ripartizione dei clandestini in Europa. Non è successo nulla. Quell'accordo è fallito: Malta si gira dall'altra parte e non soccorre nessuno, quando qualcuno arriva nelle sue acque territoriali. Con questo decreto torna l'Italia dello spreco tipo CARA di Mineo; torna l'Italia di Buzzi, che diceva che si guadagna più con gli immigrati che con la droga.

Peggiorano le procedure della magistratura, già lente e farraginose. Già ora è difficile fare un respingimento o un'espulsione e lo sarà ancora di più. inoltre, quel concetto di protezione umanitaria che non c'entra con l'asilo, che è sacrosanto e affermato nella Costituzione per chi scappa da guerre e cerca rifugio. La protezione umanitaria sarà utilizzata in maniera pretestuosa da chi si dichiarerà fintamente appartenente a questa o a quella categoria, a questo o a quello stile di vita solo per dirsi discriminato e sfuggire all'espulsione da clandestino. Riaprite alle ONG. Questo è un decreto Carola Rackete, che voleva uccidere gli appartenenti alla Guardia di finanza. *(Applausi)*. È il decreto per i trafficanti di persone, che sono il vostro modello, quelli che hanno causato più viaggi e più morti, che hanno gravi responsabilità. Noi siamo dalla parte delle vere ONG che assistono chi soffre nel mondo. Siamo contro i Leoncavallo del mare, i centri sociali del mare, che fanno una politica assurda e sbagliata, da noi mai condivisa.

Devo anche dire che la comunità internazionale dovrebbe avere più coraggio. Più volte ho detto che i fondamentalisti noti e riconosciuti andrebbero trattenuti con una legge speciale come quella che si fece in Italia ai tempi del terrorismo. Ci avete fatto caso? Appena c'è un attentato, dopo pochi minuti si conoscono la biografia, le imprese e i precedenti degli attentatori, perché erano già conosciuti e schedati. Nessuno però li ferma. Mi direte: «Ma tu li vuoi trattenere?». Sapete che cosa succede a questi attentatori? Vengono quasi tutti uccisi nei conflitti a fuoco che si determinano dopo gli attentati. Sarebbe meglio trattenerli prima, invece che lasciargli uccidere degli innocenti dopo e farli morire sulla strada, perché questo accade. C'è una pena di morte non autorizzata,

Si riducono i termini di trattenimento; si mortifica qualsiasi azione di contrasto alla clandestinità e alla circolazione di varie imbarcazioni che arrivano in Italia. Ci sono anche i rapporti internazionali. Vogliamo chiarezza dall'Egitto sulla vicenda Regeni, ci mancherebbe altro. Ma, attenzione: l'Egitto ogni anno ha 1.000 persone, tra soldati e poliziotti, che muoiono nella lotta al fondamentalismo nel Sinai e altrove. L'Egitto impedisce che milioni di persone dal Sudan e dall'Egitto stesso vadano in Libia e scappino in Italia. Verità sui casi drammatici, ma anche attenzione a non rompere rapporti. Voglio poi dire ai grillini: voi votate a seconda delle stagioni. Avete votato i decreti sicurezza con il e votate contro il decreto sicurezza nel Conte-*bis*, perché il vostro decreto è stare a galla in Parlamento e conservare il posto. *(Applausi).* Lo avete fatto anche in una vicenda che ben conosco. Quando c'è stata la vicenda Diciotti, che coinvolgeva l'allora Ministro dell'interno Salvini, eravate al Governo e avete votato giustamente a favore della relazione e delle immunità parlamentari del Senato e relatore, dicendo che il Ministro aveva agito per un interesse nazionale, nell'ambito delle sue competenze nella condivisione di Governo. Quando c'è stato il caso Gregoretti, dove il Governo era ancora più coinvolto che nel caso Diciotti, Conte ha fatto scrivere delle *mail* dal suo consigliere diplomatico Benassi al rappresentante Massari a Bruxelles, in cui diceva che o si faceva la condivisione dei clandestini o non si potevano fare altri sbarchi.

perché il vostro orizzonte è il mantenimento del posto, non una linea politica sull'immigrazione e sulla sicurezza. *(Applausi)*. Questo è un posto di lavoro - mi suggerisce il senatore Malan - non avendone altri, questa è una fortuna che vi ha colpiti. Signor Presidente, questo decreto è la resa all'immigrazione, è meno sicurezza e più clandestini, il vostro Governo è un pericolo per la salute, per i confini, per la vita quotidiana. Per questo vi diciamo no e bocciamo i vostri decreti. decreti. Avrete forse la fiducia di un Senato spaventato dal taglio dei seggi, dal crollo delle percentuali grilline, dalle verifiche poltronare di Renzi, ma non avrete la fiducia degli italiani e non avrete la nostra. Anzi, vi lasceremo votare da soli un provvedimento imposto con ottusità, senza dialogo, senza confronto, con la fiducia simultanea, senza discutere nulla. Blindate un decreto dannoso, ma se qui riuscirete ad avere un sì, avete un no nel Paese, che è già maggioranza, attraverso di noi, attraverso Forza Italia. È l'Italia della gente perbene, che dice no a voi e al vostro Governo.

Signor Presidente, farò qualche riflessione su questi decreti-legge. Teoricamente, dovrei essere il più arrabbiato perché sto pagando anche sulla mia pelle personalmente, non delegando o dimenticando, in un'aula di tribunale, l'orgoglio di aver applicato la legge, salvato vite e difeso il mio Paese. *(Applausi)*. A differenza di altri, non scappo, non dimentico, non rinnego. Ho sentito tante inesattezze, perché i numeri sono numeri. Io ricordo che, grazie a questi decreti che una parte di questa (penso ai Cinque Stelle) votò, giustamente, abbiamo dimezzato il numero dei morti e dei dispersi nel Mar Mediterraneo, quindi l'equilibrio più morti-più sbarchi è sulla vostra coscienza. *(Applausi)*. È sulla coscienza dei Ruotolo, Ci rivediamo qui fra un anno e vediamo quanto sangue sarà stato sparso nel nome della vostra presunta bontà. Più gente parte,

Io capisco che ci sia gente impegnata a prenotarsi il treno per tornare a casa, ma se, senatrice, non le interessa può uscire dall'Aula.

Gli unici che festeggeranno sono scafisti, trafficanti e sfruttatori di uomini e donne a cui questa Assemblea oggi sta facendo un regalo. ritiene. Comunque, poiché alla fine è il popolo a decidere, sarà un *referendum*, per cui a Covid esaurito cominceremo a lavorare, a cancellare questa pagina vergognosa della storia italiana. perché per arrivare in Italia bisogna avere i titoli e il permesso di arrivare in Italia, soprattutto per rispetto di chi scappa davvero dalla guerra e non va confuso con i furbetti del telefonino e per rispetto dei nostri nonni e bisnonni, che se ne sono andati dall'Italia emigrando nel resto del mondo, portando rispetto, fatica e sudore *(Applausi)*, senza che nessuno regalasse loro niente. Però, permettetemi di dire - e su questo non ci convinceremo mai - che, secondo me, è surreale. Oggi è venerdì pomeriggio. Sono le ore 16 del 18 dicembre. PD e 5 Stelle hanno certezze sui diritti degli immigrati irregolari, ma non su quelli di sessanta milioni di italiani che, ad oggi, non hanno ancora capito cosa potranno fare dalla vigilia di Natale in poi. Siete vergognosi. Siete assolutamente indegni e vergognosi. L'immigrazione non c'entra. Le indiscrezioni dicono che la soluzione del litigio...

idea un po' rossi, un po' arancioni; un po' chiusi, un po' aperti. Pare che PD, MoVimento 5 Stelle e Italia Viva,

28, 29 e 30, forse, citando il Ministro degli affari esteri, verrà permesso a qualche italiano di uscire dai confini del suo Comune, ma la mediazione Conte-Renzi pare abbia stabilito in cinquemila il numero di abitanti sopra il quale si perde questo diritto. Quindi i cittadini di Gazzaniga, in Val Seriana, in provincia di Bergamo, che sono in 5.006, non escono di casa; ugualmente quelli di Montefalco, in provincia di Perugia, quelli di Mineo, in provincia di Catania, e quelli di Recco, Borgoricco e Alberobello, perché sono in 5.000 più uno. *(Commenti)*. Capisco che questi se ne strafottano della vita degli italiani, però, se non vi interessa, uscite dall'Aula. Per voi lo stipendio a fine mese è garantito, per i baristi che devono chiudere nessuno garantisce lo stipendio.

Siamo in Parlamento. Ognuno deve poter dire quello che vuole. Dopo, interverrete voi per dire quello che volete. Senatore Santangelo, sia rispettoso nei confronti della Presidenza. Si sieda, per cortesia. Subito dopo, avrà la possibilità di esprimere il suo punto di vista. Ognuno dice la sua, ci mancherebbe altro. Prego,

a quegli imprenditori e a quei commercianti a cui Conte, il vostro Presidente del Consiglio, ha chiuso le attività per due mesi, dicendo che così almeno

o vi appellate all'incapacità di intendere e di volere? Il dubbio è questo. Vi dico però che non c'è nessun decreto al mondo che possa separare le famiglie ed evitare agli italiani di aiutare altri italiani. Nessun decreto al mondo può impedire ai genitori separati di esercitare il loro diritto. Lo dico in anticipo: siccome in silenzio, come tanti altri colleghi - immagino - e tanti altri italiani, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano e l'ultimo dell'anno, una parte delle mie giornate l'ho sempre dedicata a portare qualcosa agli ultimi ai dimenticati (una coperta *(Applausi)*, una tazza di latte caldo, un piatto di pasta, un paio di scarpe) in strada, a chi una casa non ce l'ha, il 24 e 25 dicembre esco di casa e vado ad aiutare chi ha bisogno. *(Applausi)*. Nessun decreto al mondo può impedire agli italiani di aiutare chi ha bisogno, di portare...

intollerabile tutto questo chiasso. Per cortesia, ci dev'essere rispetto reciproco, ovviamente.

per la latitanza del ministro Azzolina, da cui dipende la sorte di otto milioni di studenti di questo Paese *(Applausi)*, che non hanno ancora capito chi va a scuola e chi non va a scuola, chi sta a casa e chi non sta a casa.

chiedere ai politici se si vaccineranno, spero che non ci sia neanche un politico che scavalcherà la fila per andare a fare il fenomeno in televisione, vaccinandosi prima degli altri *(Applausi)*, perché prima vengono coloro che ne hanno bisogno. Vedremo. «Uno vale uno» anche in coda per il vaccino: non ci sono cittadini di serie A e di serie B. *(Applausi).* Sarà poi la storia a dire se avrete salvato vite o meno. Secondo me, dalla cancellazione dei decreti sicurezza ne guadagneranno la malavita organizzata e i trafficanti di esseri umani. *(Applausi).* Ricordo infatti che i trafficanti di esseri umani con il loro traffico comprano armi e droga e spero che in quest'Aula non ci sia nessuno a favore della vendita di armi (di droga non lo so, però comunque ne parleremo). Ricordo a chi vuole lo *ius soli* che con la legge attuale l'Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanza in assoluto. *(Applausi)*. Non c'è bisogno quindi di cambiare assolutamente nulla. Non vi rubo altro tempo, perché stasera perché stasera l'appuntamento non è con la lotteria degli scontrini, ma con la diretta televisiva del presidente Conte. quindi, a perdersi la diretta televisiva del presidente Conte, da Conte e da Renzi. Non penso di aver fatto cambiare idea a nessuno in questo Parlamento, ma gli italiani fuori sanno benissimo come la pensano. Spero che almeno siate coscienti del fatto che i vostri litigi, i vostri ritardi e la vostra incompetenza stanno rovinando la vita a sessanta milioni di italiani. *(Proteste)*. Spero che, prima di addormentarvi stanotte, vi facciate un esame di coscienza, perché questo Paese non merita che si tratti sulla pelle di chi, per questo Paese, ha dato tutto. Litigate su tutto, ma non sulla salute, sul lavoro e sulle famiglie dei cittadini italiani, per favore. Grazie e comunque buon Natale, sperando che la befana vi porti qualcosa di utile.

inizierei facendo i complimenti all'oratore che mi ha preceduto.

Oltretutto, abbiamo anche sentito che ha parlato degli ultimi, e questo è molto conforme all'essere il comunista padano (ce lo ricordiamo che è un comunista padano).

Ho sentito molte parole di pancia, dove però si digerisce il cibo con gli acidi, mentre noi proviamo ad affrontare il tema con il cuore e con la testa *(Applausi)*, perché questo è il classico tema da affrontare con passione e intelligenza, nonché razionalità. Eppure, una parte di quest'emiciclo, quella che sta dall'altro lato, dice sempre che fa, fa, fa. Fa? È una domanda: cosa fa? Sicuramente una cosa l'ha fatta:

che viene stigmatizzato nella sentenza della Corte costituzionale del luglio 2020, in cui si dice testualmente non viene agevolato «il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza». Non agevolare in italiano significa ostacolare

perché - e lo sapete bene - ha sempre affrontato il tema con razionalità. La nostra posizione sull'immigrazione è chiara e semplice ed è sempre stata la stessa.

hanno procurato un aumento del numero degli irregolari, da 530.000 a 600.000 in un anno. Certamente 600.000 non sono 49 milioni, ma sono comunque tanti. Abbiamo poi anche altri passaggi: si parlava del fatto che venivano controllati, ma non del modo in cui arrivava quell'80 per cento, con le imbarcazioni non controllate; ciò però serviva a fare tutta una serie di cose. Certamente siamo intervenuti e abbiamo visto che con il Governo Conte 2 il numero dei rimpatri è aumentato, anche grazie all'azione che si è concentrata negli accordi fatti pure con la Tunisia: ricorderete, colleghi, che abbiamo raddoppiato il numero degli aerei che servono a fare i rimpatri. Certo, ogni aereo può contenere un numero limitato di persone e non le famose 600.000 di qualcuno che ci disse che li avrebbe rimpatriati in un giorno, ma gli aerei da 600.000 persone non li hanno ancora inventati.

Questo abbiamo fatto: abbiamo verificato l'efficacia di un provvedimento, cercando di correggerlo, naturalmente secondo le indicazioni che ci ha dato il Presidente della Repubblica e le abrogazioni della Corte costituzionale. Dunque l'abbiamo corretto nelle parti che non erano conformi all'obiettivo. Questo è quello che abbiamo fatto ed è un percorso molto chiaro, molto semplice e molto netto. Ho sentito dire che i numeri vanno

ovvero che - purtroppo, devo dire - il numero dei morti in mare è aumentato durante il periodo in cui il senatore Salvini era Ministro.

Smettetela, fate parlare! L'ho detto prima, quando parlava il senatore Salvini, e lo stesso rispetto vale anche quando parla il senatore Cioffi, anche se esprime qualcosa sulla quale non siete d'accordo.

anch'io. Siamo una forza che è venuta in Parlamento solamente perché il sistema non funzionava. Ci stiamo lavorando con la nostra massima energia. Siamo coloro che sono entrati in Parlamento per cambiare il sistema e portare il popolo al centro dell'azione, come recita l'articolo 1

«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Mi sembra che queste siano le parole usate anche nel Vangelo e chi si richiama al cuore immacolato di Maria queste cose le dovrebbe sapere, ma evidentemente se le è scordate, perché è solo propaganda. in conclusione, quello che stigmatizziamo è l'utilizzo propagandistico del tema dell'immigrazione per... *(**Si sentono suoni

solamente per solleticare la pancia di quel popolo che quella parte dell'Assemblea vuole ignorante; noi invece non vogliamo che lo sia, perché siamo il popolo e rimarremo sempre quello che siamo: siamo entrati qua per questo solo motivo e tutti ve lo dovete ricordare!

Grazie,

E non sto parlando d'altro, cari colleghi, ma del funzionamento delle nostre istituzioni, aldilà degli schiamazzi di particolare volgarità

D'altra parte, votare la fiducia vorrebbe dire, ad esempio, signori del Governo, apprezzare o approvare questa modalità legislativa della maggioranza, divenuta normale, di uso e abuso di decreti-legge *omnibus* (accompagnati dall'immancabile voto di fiducia, per carità). E la recente invenzione, fantasiosa, sulla vicenda dei quattro decreti ristori ne è l'esempio più eclatante. Questa è una prassi consolidata, che diventa ogni giorno di più - e vi dovrebbe interessare - un monocameralismo di fatto, non normato da nessuno, ma che avviene ogni giorno per il quale troppo spesso questo Senato, colleghi, a volte anche con la vostra complicità, è ridotto a ufficio postale, dove si mette un timbro e basta. Non è una questione di Covid, la legge di bilancio è stata approvata esattamente con le stesse modalità: a scatola chiusa. Non ho la palla di vetro, ma sono sicura che anche quest'anno la legge di bilancio verrà... *(Il microfono perché non funzionano così le istituzioni, colleghi dell'opposizione, e questo non è uno stadio né un bar, ma la Camera alta di questo Paese, che meriterebbe un po' di buona educazione, oltre che di rispetto istituzionale. Credo però - e lo ripeto ai signori del Governo e agli amici dalla maggioranza - che questo sistema di legiferare debba finire.

Per questo, con il collega Richetti, mi asterrò dal Dopo aver tradito sul TAV; dopo aver tradito sul MES; il «mai col partito di Bibbiano» lo lasciamo perdere; dopo avere raccontato che mai così tanti soldi sarebbero arrivati in Italia, ma poi non trovate i soldi per risarcire i risparmiatori, gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani e le partite IVA (addirittura il piatto piange pure sul superbonus e sul *cashback*); dopo aver consentito alle multinazionali di licenziare e fare quello che vogliono, da ArcelorMittal a Whirlpool, insomma, cosa mancava all'appello dei tradimenti? I decreti sicurezza. Così, anche i taxi del mare di Di Maio li abbiamo giubilati. Se fossi in Fassino, oggi esulterei. Fassino, hai vinto! Era solo questione di tempo: il PD ha addomesticato Grillo e i grillini. Ormai i mutanti hanno compiuto la trasformazione e sono diventati un perfetto corpo del centrosinistra, un Governo europeista, amico delle banche e del sistema e avverso ai lavoratori; quei lavoratori che ora, con le modifiche di questo nuovo pacchetto, si troveranno migliaia di concorrenti sleali, immigrati, i quali accetteranno di lavorare in spregio a qualsiasi norma, salari in testa. Il PD voleva la prova d'amore e il MoVimento 5 Stelle gliel'ha data. Dopo aver negato alle famiglie di abbracciarsi per Natale, parte la rumba della finta accoglienza degli immigrati. Sotto le feste, il Viminale schiera 70.000 uomini per controllare che gli italiani facciano bene i sudditi e di contro, per controllare il traffico degli esseri umani nel Mediterraneo, vi affidate alle misericordiose ONG, i vecchi taxi del mare, a cui avete ridato di fatto il lasciapassare. E siccome l'Europa vi comanda a bacchetta, non ci sarà nessuna redistribuzione. L'ingenuità del Candido, o dell'Idiota, sta proprio nell'assecondare il gioco diabolico di chi, in nome del buonismo, sta consentendo di distruggere gli Stati, le Nazioni, la Patria, chiudendoli nella trappola dei debiti finanziari e dell'invasione dei migranti. Dall'alto il MES, i mercati, le grandi banche; dal basso, i barconi; in mezzo, gli italiani che lasciate senza lavoro, carichi di debiti e minacciati da migranti spinti a lasciare i loro Paesi dalle stesse logiche neocoloniali (vedi Macron) o dal neoliberismo, che fa leva su un senso di *pietas* che avete distorto.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

del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto,

Mininno).* Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mininno.

La prossima volta non darò più la precedenza a chi manifesta alcune necessità, perché ho dovuto riscontrare - e mi sembra un segno di mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi

che la Corte costituzionale, oggi riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta, mi ha eletto Presidente. Firmato: Giancarlo Coraggio». Complimenti al presidente Coraggio e auguri di un buon lavoro.

del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge

Signor Presidente, intervengo per una questione molto grave, perché non siamo solo in emergenza sanitaria ed economica: dal 1° gennaio entreranno in vigore ulteriori norme europee

Queste norme ferree sulla struttura e sul consolidamento finanziario rischiano veramente di fare del male alle nostre famiglie e al nostro sistema produttivo. Quindi chiedo cortesemente al Presidente se può farsi carico di comunicare insieme a noi al Governo che è necessario prendere un'iniziativa di carattere europeo affinché queste norme vengano sospese,

*(M5S)*. Signor Presidente, ci sono alcune interrogazioni parlamentari su un episodio che ritengo molto grave. C'è una banca, con sede a Roma ma interessi in Sicilia, che ha avuto a che fare con i servizi segreti, anche per operazioni inconfessabili. Banca Nuova ed è di proprietà della Banca Popolare di Vicenza, quella di Zonin, sul cui *crack* la procura di Vicenza ha chiesto la condanna a dieci anni. La banca, che ha mandato sul lastrico decine di migliaia di famiglie e di imprese, è stata protetta dalle autorità vigilanti, forse per proteggere anche gli affari segreti.

L'articolo 1 del titolo I del testo unico dei doveri del giornalista, ovvero il codice di deontologia professionale, recita: «Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie». Sto parlando di Nicola Borzi, all'epoca *reporter* del quotidiano «Il Sole 24 Ore», e di Francesco Bonazzi, de «La Verità». Ebbene, il 22 aprile del prossimo anno, Borzi e Bonazzi verranno processati per violazione del segreto di Stato. Lo ha deciso il rischiano dieci anni di galera. Questa è una storia esemplare, signor Presidente e cari colleghi, di giornalisti che trovano notizie, dunque fanno il loro lavoro e, proprio a causa di ciò, finiscono nei guai, nei tempi bui del declino della libertà di stampa, del trionfo del precariato e della sostanziale indifferenza della categoria. Borzi e Bonazzi, infatti, non sono stati difesi dall'Ordine dei giornalisti, come accade con eccellenze del nostro giornalismo come Vittorio Feltri ed Emilio Fede. Questo perché Borzi e Bonazzi non sono stati difesi da nessuno dei loro colleghi, sempre pronti ad alzare barricate per chi i fatti a volte li nasconde e li omette. In Italia, i giornalisti che fanno il proprio dovere vengono messi all'angolo, perseguitati, calunniati e denunciati, come accade, quasi settimanalmente, ai giornalisti di «Report», come accade oggi a Borzi e Bonazzi. Signor Presidente, in conclusione, ciò che dovrebbe essere una virtù viene fatto passare per colpa nel Paese alla rovescia, con onesti e servitori dello Stato perseguitati e faccendieri e pregiudicati premiati. Questo è il Paese che vogliamo? Questa è la libertà di stampa di cui ci riempiamo la bocca? Questa è la giustizia che celebriamo? Mi rivolgo a voi, cari colleghi, a tutte le senatrici e ai senatori,

ricordiamoci che, senza libertà di stampa, non c'è democrazia e che, senza conoscenza, non c'è libertà. *(Applausi)*. a chi è rimasto in Aula e anche a chi li potrà cogliere da fuori, rivolgo tanti auguri di un buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, sperando in un anno nuovo migliore. Il 28